L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei documenti VIII, nn. 9 (Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2016) e 10 (Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2017).

alla riunione dei Presidenti di Commissione, che, in base al Regolamento, in quanto Presidente della Commissione bilancio ho avuto l'onore di presiedere, ha presentato il rendiconto delle

facendo quello che molto più umilmente sto provando a fare io adesso, cominciava così: «Signor Presidente, un'opinione pubblica sempre più esigente» trent'anni fa «guarda con qualche spunto critico, che talvolta diventa acuto e pesante, il nostro lavoro... Credo che faccia parte della dignità del nostro modo di porci di fronte all'opinione pubblica la capacità di dare da un lato l'esempio di una organizzazione tendente all'eccellenza di una organizzazione tendente all'eccellenza e dall'altro l'esempio di controllabilità sia dei costi che dei moduli organizzativi». Si potrebbe dire: fare il meglio possibile con il massimo di risparmio delle risorse pubbliche possibile. Poi, qualche passaggio dopo, aggiungeva: «Non possiamo non prendere atto che negli ultimi dieci anni,

negli anni Ottanta in cui la spesa del Senato aumentò del 36 per cento rispetto all'anno prima: la media era del 25 «e che soltanto dal 1988 (cioè dall'anno prima) noi stiamo muovendoci intorno al 10 per cento di incremento della spesa». ma è troppo interessante da leggere oggi, che misura l'ampiezza del percorso per abbiamo fatto.

l'età dell'oro non è mai esistita, e forse quell'età era dell'oro nel senso che si spendeva e si sprecava. Per fortuna, c'erano anche uomini come Nino Andreatta che si battevano per un uso più oculato delle risorse. I senatori Questori saranno molto più puntuali di me, però ci stiamo muovendo su tutt'altro ordine di grandezze: il consuntivo del Senato 2012 aveva chiuso a 520 milioni euro; oggi discutiamo di un rendiconto 2016, quello che ci è stato presentato dai senatori Questori, che riduce le risorse utilizzate dal Senato a 492 milioni di euro. per cento di aumento che Andreatta considerava un grande risultato! Qui c'è un taglio del bilancio nominale, quindi una riduzione secca di risorse disponibili: 28 milioni di euro in meno nell'arco della legislatura, ogni anno; una riduzione del bilancio in termini nominali: un risultato lusinghiero per l'Amministrazione del Senato, ovviamente per la Presidenza del Senato, per i senatori Questori, per il Segretario Generale e per tutta la macchina del Senato che può presentarsi con un bilancio di tutto rispetto. Possiamo dire ai cittadini italiani che stiamo facendo quello che tutto lo Stato dovrebbe fare - naturalmente, sappiamo che il bilancio dello Stato è molto più complesso - ovvero fare meglio e cercare di svolgere al meglio la nostra funzione imparando a spendere di meno. Questo è un pallino per chi ha, *pro tempore*, il ruolo di guidare la Commissione bilancio, ma dovrebbe essere un assillo che ci coinvolge tutti; certamente ci ha coinvolto tutti come Senato della Repubblica. Oggi possiamo dire ai nostri concittadini che il Senato costa certamente meno di quanto costava all'inizio di questa legislatura; costa di meno non solo in termini reali, ma anche in termini nominali, e questo credo che sia un risultato di grande importanza. Detto ciò, non siamo qui soltanto per farci i complimenti - anche se ogni tanto darci un po' di incoraggiamento sul lavoro positivo che stiamo svolgendo credo che sia utile - ma siamo qui anche per riflettere sulle cose che vanno ancora affrontate. Se guardiamo le tabelle presentate nel rendiconto, dopo la prima tabella che misura il percorso che abbiamo compiuto,

la spesa di funzionamento generale e la spesa previdenziale. Quest'ultima è ancora il grande *handicap* del bilancio del Senato, sul quale peraltro c'è una piccola notazione positiva, che poi farò presente.

il 45 per cento) è la spesa previdenziale, sommando la spesa previdenziale per gli ex senatori e quella per egli ex dipendenti del Senato.

immaginando percorsi lunghi. La tabella n. 7 del rendiconto ci dice alcune cose che è importante sapere. La prima è che

Naturalmente la spesa per i vitalizi ha un andamento sinusoidale, perché si impenna all'inizio della legislatura, quando un numero consistente di senatori non

Ci sarebbe bisogno di un approfondimento più particolareggiato, ma credo che una parte di questa tendenza al risparmio sia dovuta alle riforme che sono state fatte negli anni passati: mi riferisco a quelle di dieci anni fa, in modo particolare, che hanno ridotto il rendimento, sia pur del sistema ancora retributivo, e hanno aumentato in maniera significativa l'età minima per poter accedere all'allora vitalizio. Da ultimo, nel 2012 vi è stata la riforma la riforma che ha introdotto il sistema contributivo anche per gli ex senatori. Più problematico, invece, a me pare il quadro sulla questione dei nostri grandi e fondamentali collaboratori, che sono i dipendenti del Senato, senza i quali il nostro lavoro sarebbe impossibile, ai quali quindi va tutta la nostra riconoscenza, tutta la nostra stima e, per chi è più vecchio del bosco, come il sottoscritto, anche un po' di affetto, perché sono persone con le quali lavoriamo gomito a gomito da tanto tempo. Vi è una caduta abbastanza rapida della spesa per i dipendenti in servizio, che, naturalmente, da un certo punto di vista, rappresenta un risparmio, ma che, da un altro punto di vista, sta arrivando ai limiti del depauperamento della nostra struttura. C'è quindi da fare una riflessione su questo: fino a che punto è immaginabile andare avanti con questo *trend* senza compromettere la funzionalità dei servizi essenziali del Senato? è un aumento molto forte della spesa per le prestazioni pensionistiche per questi nostri collaboratori: naturalmente chi va in pensione esce dal capitolo «Personale dipendente in servizio» ed entra nel capitolo di spesa «Personale in quiescenza»; e la crescita della voce «Personale in quiescenza», come vedete dalla tabella n. 7, è molto elevata. Non è questa la sede per approfondire la questione, ma certamente occorre trovare una soluzione rispettosa di ciò che è stato maturato, delle carriere

si debba spingere con forza, come so che il Consiglio di Presidenza sta facendo e ha fatto da molto tempo a questa parte, verso il ruolo unico del personale di Camera e Senato, in modo da garantire un'ottimale distribuzione delle risorse tra i servizi comuni: tutto ciò che può essere messo in comune, come so che

dal punto di vista delle previsioni macroeconomiche e, quindi, dal punto di vista delle manovre finanziarie che il Parlamento deve approvare. Voi sapete che si parlava da tanti anni di istituire un'autorità del genere, genere, che, poi, è stata fortemente caldeggiata in sede europea, dopo le vicende della crisi greca, che in parte furono dovute proprio a a bilanci non affidabili; pertanto, l'affidabilità del bilancio pubblico è diventata un elemento essenziale anche nelle relazioni europee. Si è, quindi, costituito l'Ufficio parlamentare del bilancio,

il fallo, richiamando il Governo alla correttezza delle previsioni macroeconomiche per il 2017. L'Ufficio parlamentare di bilancio non validò, nell'autunno dell'anno scorso, le previsioni di crescita del Governo per il 2017, in qualche modo costringendolo a rivederle.

credo che sia stata una vittoria del Parlamento il fatto che, grazie a questa struttura che abbiamo istituito e voluto che fosse nel Parlamento e non al di fuori, il Governo è stato costretto a tornare alle Camere, aggiustando i conti così

i Capigruppo della Commissione bilancio, naturalmente avendo prima sentito e concordato con i senatori Questori, la Presidenza e la Segreteria generale, affinché si risolva il problema delle strutture di Questo è il quadro complessivo, così come è stato affrontato nella riunione dei Presidenti di Commissione. Come sempre, la discussione sul bilancio è anche un'utile opportunità per ragionare sul nostro modo di lavorare. Alcuni colleghi hanno rilanciato la questione annosa della ripartizione dei compiti tra Assemblea e Commissioni, e Commissioni, che certamente è uno dei punti nevralgici del nostro lavoro e sono tanti i temi sul funzionamento di quest'Assemblea. Un Parlamento vivo - noi tutti crediamo in un Parlamento come

2017, oltre al bilancio triennale 2017-2019. In questo mio breve intervento farò una veloce disamina dei documenti contabili, illustrandone le cifre principali che rappresentano i frutti sul fronte di contenimento della spesa, raggiunti dagli organi di direzione politica di questo ramo del Parlamento. Per maggiori dettagli, come è ovvio, vi rimando ai documenti contabili allegati al Resoconto di seduta.

Credo che questo sia un aspetto veramente fondamentale ed importante. Rispetto al 2015, sia la spesa di funzionamento, previdenziale scendono sotto livelli che non si sono mai raggiunti e teniamo conto che nei bilanci della pubblica amministrazione, come in quelli di tutte le aziende, questa spesa non è mai considerata all'interno del bilancio stesso.

Per quanto riguarda il trattamento delle cariche interne, da subito nel 2013, appena insediato, il Presidente del Senato ha voluto, nella prima riunione del Consiglio di Presidenza, operare

importante. Questo ci ha portati anche alla dematerializzazione degli atti parlamentari: ben 18.659 atti sono stati pubblicati in formato digitale, mentre altri 153.000 atti sono nell'archivio digitale del Senato, con un risparmio di ulteriori

Ricordo anche l'attenzione che abbiamo voluto dare al Senato stesso, con la ripresa delle manutenzioni al nostro interno: dalle piccole alle grandi manutenzioni che abbiamo visto, sia

Altrettanto, in questa legislatura noi abbiamo realizzato un risparmio di 188,11 milioni di euro per il funzionamento del Senato. Quindi, lo Stato in cinque anni spende 188 milioni di euro in meno. Questo è un aspetto veramente importante. 108 milioni di euro di minore dotazione da parte dello Stato che, se calcoliamo anche l'aspetto reale, in termini reali, della dotazione, ci ci porta al minimo storico rispetto a tutti gli anni precedenti; 80 milioni di euro di somme restituite alle casse pubbliche e, quindi, allo Stato stesso. stesso. Il costo del Senato è diminuito, rispetto alla spesa statale, dallo 0,083 allo 0,059. Praticamente, per ogni mille euro che lo Stato spende, il Senato spende 0,59 centesimi. Questo è un altro degli aspetti importanti che prima anche il presidente Tonini citava nel percorso del risparmio e dell'attenzione che abbiamo voluto dare in questi anni al Senato stesso. Il Senato si poggia su tre pilastri: il personale, quello di noi senatori e quello dei servizi. Parto da subito dai senatori che, anche in questi giorni come in questi anni, sono sempre più vituperati per le spese e per altre questioni. Abbiamo ottenuto un contenimento dell'indennità e delle competenze accessorie di 37,2 milioni di euro. Dal 2001 al 2017 il rapporto tra la spesa per le indennità dei senatori e il bilancio del Senato si è dimezzato: si passa dal 19 per cento al 10 cento. Questo è un aspetto importante da ribadire in quest'Aula. Si aggiunge a questo, poi, anche il contributo di solidarietà del 2014-2016 che porta un risparmio di ulteriori 17 milioni di euro. un altro dato positivo del nostro percorso di questi anni. Altro pilastro fondamentale per il Senato, ma credo sia così per tutte le istituzioni, è quello del personale.

nella collaborazione con la Camera rispetto al ruolo unico del personale stesso, nelle integrazioni funzionali che abbiamo fatto per la rimessa in moto, tra i due rami del Parlamento, anche di

e tutta una serie di altre gare in corso di definizione, come la prestampa, la rassegna stampa, il monitoraggio radiotelevisivo, il nuovo sistema di ripresa video dell'Aula, la cassa del Senato, il canale satellitare.

Tutte queste ulteriori gare e riduzioni possono indurci a effettuare una stima prudenziale per il 2017 di 16 milioni di euro di ulteriori risparmi e altri possono arrivare con l'integrazione tra Camera e Senato.

Queste integrazioni funzionali hanno già prodotto dei poli parlamentari, dove si sono messi assieme più uffici, quali i servizi sanitari, i servizi informatici, i servizi di documentazione, con l'implementazione del già esistente polo bibliotecario e degli archivi storici. previsto anche tutto uno schema procedurale per le gare comuni, da fare tra Camera e Senato. Già alcune gare sono state espletate assieme da Camera e Senato: parlo della gestione dei servizi informatici, di assistenza all'utenza, della prestampa e della rassegna stampa e del canale

cui vorrei rivolgere un grazie particolare per il lavoro, l'assistenza e l'aiuto che ci danno anche all'interno di questa Aula.

la valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche. Valutare le politiche pubbliche non significa entrare nel merito

capire quali sono gli effetti reali delle leggi e dei regolamenti che il Governo e il Parlamento hanno deliberato o hanno in previsione di deliberare. Serve quindi a capire se gli effetti che si producono a livello sociale ed economico economico dipendono veramente da quella specifica politica oppure no. All'estero, soprattutto nei Paesi di tradizione anglosassone, la valutazione la valutazione è una prassi ormai consolidata, che risale al secolo scorso. La Francia e il Marocco l'hanno addirittura prevista nella loro Costituzione. Per l'Italia è una strada nuova La valutazione, infatti, richiede uno sforzo non comune. È un insieme di tecniche molto complicate che richiedono uno sforzo d'apprendimento e di approfondimento. Il Senato, dopo due anni di esperienza con altre realtà europee e internazionali, ma soprattutto dopo due anni molto intensi di preparazione del proprio personale, è arrivato a un livello di competenza nel campo

in cui si spazia dalla questione carceraria all'analisi fiscale ad altre tematiche (vi lascio la sorpresa). la strada da percorrere è ancora lunga per riuscire a coprire tutti i campi e tutti i settori necessari per il Parlamento, affinché l'azione del Governo sia efficacemente controllata da parte di chi è stato eletto dai cittadini. Il Senato, tuttavia, è già oggi in grado di percorrere, insieme ad altre istituzioni prestigiose in Europa e nel mondo, delle strade finora inedite per il nostro Paese. Va quindi dato atto che, grazie al Presidente e al supporto del Collegio dei senatori Questori, l'Amministrazione è riuscita, con umiltà ma anche con grande determinazione e - lo vorrei ribadire - a costo zero, a centrare l'obiettivo. Un ringraziamento va a tutto il personale, che si è prodigato con entusiasmo su questo progetto innovativo e in certi momenti anche faticoso. L'obiettivo riguarda tutti noi: tutti noi: valutare se i soldi dei cittadini sono stati ben spesi, rendere più efficaci le nostre leggi e non ripetere gli errori del passato. *(Applausi

Come lei sa, le Commissioni esteri e difesa si stanno per riunire per poter esprimere il loro voto in relazione alla risoluzione che discuteremo domani in Aula

in un orario ragionevole, di convocare le nostre due Commissioni, naturalmente compatibilmente con il

di riunione delle Commissioni congiunte esteri e difesa di Camera e Senato, hanno chiesto di poter avere copia della lettera con cui il Governo libico richiede l'intervento dell'Italia. È stato detto che sarebbe stata resa disponibile ai soli componenti del Copasir, a partire dalle 17. Quindi è evidente che, nella valutazione complessiva dei Gruppi,

Siamo d'accordo che non prima delle 19 noi autorizzeremo la possibilità di convocare

Presidente, mi sembra che il percorso che lei ha indicato sia quello che consente di lavorare in un certo modo. L'unica cosa che non ho capito dell'intervento del collega Fornaro è il riferimento alla famosa lettera mandata dal Governo libico Noi riteniamo - ne parlavo con il collega Divina, che ci rappresenta in Commissione difesa - che non debba essere un rapporto sulla conoscenza della lettera riguardante l'elemento fiduciario dei rappresentanti dei Gruppi: deve esserci un momento comune, magari segretato, con tutto quello che si può fare all'interno delle due Commissioni, dove qualcuno riferisce il contenuto della lettera. Lo dice un Gruppo che ha una rappresentanza peraltro qualificata all'interno del Copasir: ci sembra che questo sia il percorso migliore, cioè che venga segretata la seduta delle due Commissioni riunite e che in quella sede qualcuno qualificato riferisca sul contenuto della lettera.

particolarmente importante del Governo libico. Voglio però far notare che il Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE non ha nessun rappresentante all'interno del Copasir; noi saremmo quindi esclusi da una presa

ci sia qualcuno, componente del Copasir, che riferisca nelle Commissioni riunite, segretando chiaramente la seduta. Mi pare che attraverso questo sistema si possa avere la conoscenza, mantenendo la segretezza. È un modo per conciliare le due esigenze.

G28 si sposa benissimo con il concetto di trasparenza, perché con esso chiediamo che il trattamento dei senatori

la nostra richiesta di urgenza sul disegno di legge per l'abolizione dei vitalizi, addirittura appellandosi e portando ad esempio quello che accade nel Comune di Roma.

condannati in via definitiva per capire quale sia il bisogno reale del Paese e le necessità dei cittadini non c'è bisogno di far spendere allo Stato quasi 800 milioni di euro per un *referendum* costituzionale totalmente inutile; non c'è bisogno di far spendere centinaia di milioni di euro ai palazzi di Senato e Camera per fare una legge elettorale che, secondo voi, ci avrebbe copiato tutta Europa e che invece non abbiamo mai applicato. Per fare le cose in maniera equa e onesta verso

caro presidente Zanda, visto che le sta così a cuore il risultato del *referendum* - soltanto questo valore è ben superiore ai risparmi che ci avevate fatto credere che avremmo ottenuto a valle del*referendum* del 4 dicembre. Quindi, già solo per questo motivo dovreste essere d'accordo, perché andiamo ben oltre quei risparmi ai quali avevate l'auspicio di arrivare. Detto questo, che cosa chiediamo sostanzialmente con questi tre ordini del giorno, tutti In particolare, con il G18 chiediamo di disporre la cessazione dell'erogazione di vitalizi e pensioni a favore dei senatori cessati dal mandato, ivi compresi quelli di reversibilità, prevedendo la restituzione della somma corrispondente alle somme trattenute a titolo di contributi, detratti dagli importi già corrisposti, sotto forma di assegno vitalizio o pensione. Con l'ordine del giorno G22 G22 impegniamo il Collegio dei senatori Questori e il Consiglio di Presidenza

l'importo dei vitalizi a favore dei senatori cessati dal mandato, ivi compresi quelli di reversibilità, non superi tre volte l'importo del trattamento minimo annuo individuale. Qui potremmo riagganciarci al discorso fatto stamattina da un

sinceramente in questo momento, stante il fatto che oltre 8 milioni di cittadini italiani vivono al di sotto della soglia di povertà, considerare una pensione da 3.000-4.000 euro come una pensione d'oro credo sia semplicemente un esercizio stilistico: non prendiamoci in giro.

della società che chiede sacrifici a un numero così grande di italiani, probabilmente dovremmo essere i primi a dare l'esempio e a dimostrare che siamo in grado di fare ciò che, tra l'altro, non possiamo neanche chiamare «sacrifici».

condanne o coinvolti in reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, in base alla delibera del Consiglio di Presidenza del 7 maggio 2015, chiediamo di prevedere delle modifiche: ad esempio l'introduzione del reato di abuso d'ufficio nel novero di quelli la cui condanna definitiva inibisce la riscossione del vitalizio parlamentare; la cessazione del vitalizio parlamentare per i soggetti condannati in via definitiva a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, di quattro anni; dell'articolo 1, comma 4, riguardante i familiari superstiti di parlamentari condannati, deceduti prima dell'entrata in vigore della delibera. Questo sostanzialmente è ciò che chiediamo con i nostri ordini del giorno. Termino la mia illustrazione facendo una considerazione generale e richiamandomi ancora a quanto affermato dal senatore Zanda questa mattina sul concetto di vitalizio. Ripeto, questa mattina parlavamo dei vitalizi in generale, adesso siamo obbligati a farlo soltanto su farlo soltanto su quelli legati al Senato. Caro senatore Zanda, probabilmente noi saremo anche il popolo della democrazia diretta e pensiamo di attribuire un valore estremamente importante a un clic, però c'è una differenza fondamentale fra noi e voi: voi continuate imperterriti ad accedere ai finanziamenti dei cittadini, quindi a usare i soldi dei cittadini per fare i vostri interessi e le vostre autoreferenzialità; invece i nostri clic sono totalmente gratuiti e noi non chiediamo neanche un centesimo ai cittadini italiani. Ed è per questo che noi possiamo uscire da questo Palazzo e camminare a testa alta. I nostri portavoce possono andare in giro senza scorta perché non abbiamo nulla da temere.

secondo me, sono importanti per tutti e comunque a me molto cari. Il primo è una richiesta di maggiore trasparenza nei bilanci, era stata avanzata anche l'anno scorso

Questa Istituzione per fortuna vive e sopravvive nonostante le persone che la interpretano, da quando è stata fondata fino a quando avrà la fortuna di sopravvivere. Sarebbe importante, credo, che ciascuno di noi si rendesse conto di essere solo un interprete transitorio di un'Istituzione che ha una dignità che, per fortuna, prevale sulla capacità del singolo di far vedere un minimo di dignità (a volte, veramente un minimo). Il tema del denaro è sicuramente rilevante, ma credo che sia anche importante dare fuori di qui un messaggio molto chiaro. La lista dei risparmi che ha fatto il senatore Questore De Poli le richieste, anche insistenti, dei colleghi che mi hanno preceduta, credo che debbano essere affermate tenendo sempre presente che c'è un contenuto che deve essere alto. Qui il tema non è solo quello del risparmio degli spiccioli; qui il tema più rilevante è dare dimostrazione, con trasparenza, di quanto si è speso, di come lo si è speso e del risultato che si ottiene con questa spesa. Faccio un esempio. Parlando di formazione e aggiornamento del personale ho notato che quest'anno vi è un grande aumento rispetto sia alla previsione scorsi, sia alle cifre spese gli anni scorsi. Da insegnante, non posso che rallegrarmi per il fatto che si investa sulla formazione del personale, soprattutto quando la formazione del personale della categoria di cui faccio parte, gli insegnanti, generalmente viene fatta in autoformazione

perché la trasparenza non è un'arma che viene imbracciata da qualcuno e rivolta contro gli altri; la trasparenza deve essere vissuta e percepita come una garanzia per tutti,

Credo che la trasparenza sia nell'interesse di tutti e sia anche uno strumento importante per dare dignità al denaro che abbiamo speso, soprattutto in relazione all'altezza delle motivazioni per cui è stato speso. Infatti, anche se risparmio e riduco le mie spese del 50 per cento, ma spendo il denaro in una percezione, che purtroppo i cittadini hanno, di inutilità inutilità di questa Istituzione, potrò anche risparmiare molto, ma non avrò ottenuto quello che volevo ottenere. Signor Presidente, le chiedo solo altri due minuti

Presidente, lo sa bene: un giorno le è arrivata una lettera che le comunicava che io non facevo più parte del Gruppo con il quale ero stata eletta. Intanto, pretenderei

quanto alla relazione che c'è tra il parlamentare che è stato eletto e il contesto nel quale è stato eletto. Io sono fortunata, perché di fatto il Movimento 5 Stelle nella mia Regione

della scuola eletta nel Partito Democratico non avrei potuto minimamente riconoscermi in come il Partito Democratico ha portato avanti la riforma della scuola e, forse, legittimamente, avrei reso un miglior servizio ai miei elettori uscendo da quel Gruppo e andando altrove e, particolarmente, nel Gruppo Misto, che in questa legislatura è diventato, di fatto, il luogo che ha raccolto testimoni di coerenza, oltre a quelli che vengono In un ordine del giorno chiedo che l'Istituzione si faccia carico trovando qualche soluzione, che potrebbe anche essere, ad esempio, quella adottata dal Parlamento europeo, che assume direttamente quattro soggetti per ciascuno di coloro che sono i rappresentanti, garantendo così che quel singolo possa avere la facoltà di lavorare a prescindere da qualunque vincolo con il proprio Gruppo, al quale, a un certo punto, anche per ragioni indipendenti dalla sua volontà, potrebbe non potere o non volere appartenere più. Quindi, io chiedo che venga trovata una soluzione per garantire, in sostanza, l'efficacia dell'articolo 67 della Costituzione.

che serve a coprire le spese d'ufficio e dei dipendenti.

un lavoro a persone che vogliono collaborare nell'attività politica. Come è noto a tutti quanti noi, parte dei componenti di questo importante consesso rendicontano versando

a incrementare ciò che serve a far vivere il senatore, oltre all'indennità che già gli spetta.

l'esame del progetto di bilancio interno e del rendiconto costituisce un appuntamento importante per la vita della nostra istituzione»: con queste parole iniziavo il mio intervento sui documenti di bilancio interno nel settembre 2014

dopo che il *referendum* del 4 dicembre dello scorso anno ha confermato il bicameralismo così come è stato definito dai nostri Padri costituenti. Va apprezzata l'attenta opera del Collegio dei Questori, del Presidente, dell'Amministrazione che si è sviluppata in questi anni realizzando ottimi risultati nella gestione delle spese, avendo però anche uno sguardo attento sugli effetti che sarebbero potuti derivare dall'approvazione definitiva della riforma costituzionale.

Il risultato è altamente positivo se si pensa che è stato conseguito senza alcuna flessione nel livello dei servizi erogati nei diversi settori dell'Amministrazione. dell'Amministrazione. Il Presidente, il Collegio dei Questori e l'Amministrazione hanno gestito le complesse funzioni esistenti avendo uno sguardo ai possibili effetti che su queste avrebbe avuto la riforma costituzionale. Da questo punto di vista, va espresso il più vivo apprezzamento per i seminari di aggiornamento professionale aperti a tutti i dipendenti, indipendentemente dal ruolo rivestito, e per essere stato il Senato capofila nella promozione, con la collaborazione di istituzioni prestigiose come l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Istituto per la ricerca valutativa sulle politiche pubbliche di Trento e l'Associazione per lo sviluppo della valutazione e l'analisi delle politiche

Anche in tal modo il Senato si è preparato rispetto agli eventuali nuovi compiti che gli sarebbero stati assegnati, operando, nel contempo, nella direzione di un ulteriore consolidamento su materie di stringente attualità della preparazione dei dipendenti, confermandone gli elevati *standard*. Come ho detto prima, questo è il primo bilancio del Senato riconfermato nel modello costituzionale del 1948 ed è quindi l'occasione per una riflessione complessiva che conduca alla definizione in prospettiva di direttrici coerenti con quel modello, così come è stato fatto nel passato. Dal punto di vista qualitativo sono stati conseguiti risultati positivi sul versante, tra l'altro, della comunicazione e del monitoraggio delle fonti di informazione; del contenimento, del consumo e della fornitura di energia esclusivamente da fonti rinnovabili; della lotta allo spreco alimentare e delle infrastrutture informatiche, come ricordato nella relazione del senatore De Poli. L'analisi che ho prima brevemente tracciato delle somme iscritte nel bilancio interno, da un lato, testimonia l'impegno del Senato a proseguire nella politica di contenimento della spesa in un quadro economico che solo ora presenta qualche dato incoraggiante e, dall'altro, dà una risposta concreta alle ricorrenti polemiche sui costi di questo ramo del Parlamento e, più in generale, degli organi costituzionali. È tuttavia necessario rifuggire da qualsiasi logica che affronti l'argomento del funzionamento delle istituzioni in termini di semplici costi. L'anticasta continua a puntare il dito inquisitore sui costi delle istituzioni rappresentative ed è giunto il momento di chiedersi se ciò che il Paese deve continuare a guardare sono i costi della democrazia rappresentativa o o se, piuttosto, il vero obiettivo di quell'indice inquisitore non sia il superamento stesso del modello di democrazia rappresentativa previsto dal nostro ordinamento. Per parte mia, continuo a essere profondamente convinto che questo modello costituisca l'unico strumento per la realizzazione dei principi democratici anche in una società complessa come la nostra e che il rispetto delle regole del gioco o - come sono state anche chiamate - degli "universali procedurali" sia ineludibile. I dati finanziari in precedenza descritti appartengono al patrimonio dei risultati quantitativi e qualitativi che il Presidente, i Questori e l'Amministrazione hanno conseguito in questa legislatura. Ma il fatto che questo sia il primo bilancio del Senato dopo la conferma del suo assetto con il *referendum* del dicembre scorso ci deve indurre a individuare le linee guida che - a mio avviso - dovranno essere seguite nel futuro per consolidare ancora di più il ruolo di questo ramo del Parlamento. Per quanto riguarda il trattamento dei senatori, mi sembra di poter dire che i risultati di contenimento della spesa conseguiti in questo settore siano rilevanti e, d'altra parte, non dimentichiamo che - come ebbe a chiarire già anni fa la Commissione Giovannini - il costo complessivo a titolo di trattamento economico delle Assemblee dei Paesi europei con il PIL più elevato è superiore a quello sostenuto per i parlamentari italiani. Le questioni relative al trattamento economico dei senatori devono - a mio avviso - essere affrontate con animo scevro da pregiudizi, facendo bene attenzione a distinguere ciò che è privilegio da ciò che è invece semplice espressione di prerogative. Non dimentichiamo che l'indennità è un istituto costituzionalmente previsto: l'articolo 69 della Costituzione stabilisce, infatti, il carattere non gratuito del mandato parlamentare e questa disposizione è il modo con il quale viene data attuazione al principio democratico per cui tutti i cittadini devono poter accedere alle cariche elettive in posizione di eguaglianza, come previsto dall'articolo 51 della Carta fondamentale. Una attenzione particolare va poi posta al tema dei dipendenti del Senato. Si tratta di personale che, a ogni livello, ha superato concorsi estremamente severi, aperti a tutti e ai quali ciascuno era libero di partecipare, e che hanno consentito alla nostra Istituzione di assicurarsi le migliori energie tra quanti di anno in anno si affacciavano al mondo del lavoro. un personale chiamato a svolgere le sue funzioni al servizio dell'Istituzione con professionalità, competenza, serietà e dedizione, senza orario e al di fuori di qualsiasi prevedibilità, come solitamente è la nostra attività parlamentare, fatta di persone, donne e uomini, che ci sono professionalmente vicine. Ed è quindi questa l'occasione per rivolgere un convinto, sentito ringraziamento a tutti i dipendenti. È dunque necessario adottare le opportune misure per preservare questo patrimonio di eccellenza. Nel maggio scorso le Amministrazioni del Senato e della Camera hanno ricevuto mandato dal Consiglio di Presidenza del Senato e dall'Ufficio di Presidenza della Camera - come ha appunto rilevato il senatore De Poli - di sottoscrivere protocolli d'intesa concernenti il polo della documentazione parlamentare; un *addendum* al polo bibliotecario, già sperimentati positivamente; il polo informatico parlamentare; il polo dei servizi sanitari; la collaborazione per gli archivi storici. Sono state quindi poste le premesse per una sempre più completa integrazione delle attività e delle risorse e ritengo sia quindi opportuno procedere con determinazione lungo le direttrici indicate dai protocolli. Infine, un problema centrale per il funzionamento della nostra Istituzione è quello del reclutamento del personale. Le Amministrazioni dei due rami del Parlamento devono operare per concludere l'attività istruttoria diretta ad attuare tutti gli adempimenti previsti dall'accordo istitutivo del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, ciò al fine di riattivare la leva del reclutamento. Al fine di poter conseguire quest'obiettivo, sarà anche necessario definire eventuali procedure concorsuali comuni. L'attivazione della leva concorsuale riveste in questo momento particolare rilievo, poiché negli ultimi anni si è registrato un significativo decremento del numero dei dipendenti del Senato. Ed è questo un dato al quale bisogna porre rimedio nel più breve tempo possibile. Auspico che le decisioni che saranno adottate in materia nel Consiglio di Presidenza siano in linea con l'obiettivo di continuare a garantire professionalità di eccellenza e di non mutare continuamente il quadro di riferimento dei trattamenti economici che causa sconcerto e disaffezione. È necessario invece assicurare stabilità a chi, partecipando ad un concorso per l'accesso alla carriera presso il Senato, ne ha anche scelto il trattamento giuridico ed economico e non può vedere successivamente conculcati i diritti acquisiti; ciò, d'altra parte, in conformità agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale. Ricordiamo sempre che su di noi grava la responsabilità di assicurare al Senato, riconfermato nella sua struttura e nelle sue funzioni, quel patrimonio di conoscenze e di professionalità costituito dal personale. Non si può pensare di demolire ciò che è stato realizzato da chi ci ha preceduto, ma si deve garantire continuità all'operare dell'Istituzione. Quali che saranno gli obiettivi che la politica intenderà perseguire sulla base del pronunciamento degli elettori, dovrà sempre esservi un apparato amministrativo che consenta ai senatori di conseguirli nel rispetto delle regole procedurali che essi stessi si danno nell'ambito dell'autonomia regolamentare costituzionalmente sancita. qui l'importanza di quell'apparato che merita tutto il nostro rispetto e la nostra considerazione. Prima di concludere, signor Presidente, desidero rinnovare il mio ringraziamento ai senatori Questori per il non facile lavoro svolto in questi anni, che ha consentito di conseguire importanti risultati, e al personale tutto, dal Segretario Generale, ai Vice Segretari Generali, agli assistenti parlamentari, per il lavoro che quotidianamente svolgono al nostro fianco con eccellente preparazione e spirito istituzionale. Per tutte le motivazioni che ho illustrato preannuncio che il mio Gruppo voterà a favore dei documenti di bilancio al nostro esame.

Questori a deliberare affinché la totalità delle spese effettuate con le risorse percepite a titolo di «rimborso delle spese per l'esercizio del mandato» sia soggetta a sistematica e puntuale rendicontazione

si conferisca un significato concreto: il rimborso è quello che mi viene restituito una volta che do la prova di aver anticipato delle somme (questa definizione ricorda la trappola semantica dei rimborsi elettorali dei partiti, ma questo è un altro ragionamento)». Noi proponiamo che l'intera somma di 4.180 euro mensili sia oggetto di rendicontazione e di rimborso successivo.

prevede la restituzione da parte del senatore della parte di rimborso spese non utilizzata. Siccome siamo previdenti e sappiamo che è difficile sfilarvi anche un centesimo dalle tasche, abbiamo previsto un altro ordine del giorno che non prevede alcuna restituzione. State tranquilli: anche se avanzano dei soldi, basta rendicontarli. Non c'è alcun populismo. C'è solo la volontà di rendere trasparenti tutte le spese, perché parliamo di ben 2.090 euro, che oggi sono di fatto uno stipendio aggiuntivo in nero per ogni senatore. soltanto la rendicontazione per fare in modo che tutti i cittadini sappiano cosa si fa con queste somme.

del giorno G11 riguarda l'eliminazione della rimborsabilità delle erogazioni liberali

che ci viene data dal Senato della Repubblica, deve essere rendicontata al Senato almeno al 50

al mio partito politico, sto facendo un qualcosa che non riguarda l'esercizio del mandato. Si tratta di una mia erogazione spontanea e liberale che voglio fare alla mia forza politica e, quindi, è un atto personale che non rientra nell'esercizio del mandato, ossia di quel mandato che è stato dato dagli elettori.

chiediamo semplicemente di eliminare dalle voci di spesa ammissibili ai fini del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato le somme versate dai senatori ai soggetti politici, sia a titolo di erogazione liberale che quale corrispettivo o rimborso della fornitura di servizi o prestazioni ricevute.

al corrispettivo o rimborso della fornitura di servizi o prestazioni, ma vorrei lasciare l'eliminazione riferita all'erogazione liberale. L'ordine L'ordine del giorno G21 riguarda l'applicazione del metodo contributivo ai vitalizi parlamentari. Ovviamente è materia che oggi avete ritenuto non essere urgente;

a tutte quelle somme. In verità è già stato chiarito più volte che i vitalizi non si configurano come pensione, ma sono qualcosa di integrativo che non ha assolutamente tale connotazione. Noi, quindi, chiediamo semplicemente che il vitalizio

Presidente, sono quattro anni che in quest'Aula sui provvedimenti importanti, quelli che potrebbero essere veramente di aiuto ai cittadini, ci sentiamo rispondere che non c'è la disponibilità economica per poterli approvare: c'è la *spending review*, ci sono le spese c'è da rispettare quello che ci chiede l'Europa. Così dite solitamente quando non avete motivazioni adeguate. Secondo voi, nel nostro Paese non ci sono sufficienti risorse per offrire un sostegno concreto alle Forze dell'ordine.

Non ci sono sufficienti risorse economiche per mettere in sicurezza gli edifici scolastici che crollano e sono costretti a chiudere perché non a norma, come dimostra quello che sta accadendo nella Provincia di Caserta, in dissesto finanziario anche grazie alla scellerata legge Delrio, e che ha visto chiudere già diversi istituti scolastici. Dobbiamo comunque ringraziare Dio che non ci sono state vittime, visti i crolli frequenti dei tetti delle scuole. Non ci sono risorse economiche adeguate per le bonifiche delle aree inquinate che mettono a rischio la salute dei cittadini; peraltro, tale inquinamento è spesso causato da aziende a cui sono state - per così dire - rilasciate con troppa facilità le relative autorizzazioni, grazie anche ad alcuni dei vostri referenti politici locali e a enti troppo compiacenti. Non ci sono risorse per la manutenzione dei beni artistici e archeologici che ci invidiano in tutto il mondo e che qui noi lasciamo marcire come se fossero beni di scarto senza alcun valore.

Eppure, chissà come mai, i soldi per le banche li avete trovati. La settimana scorsa avete semplicemente regalato alle banche 17 miliardi di euro, ovviamente a discapito dei risparmiatori italiani. Ma, certamente, cosa vuoi che importi al Parlamento che cittadini disperati abbiano perso i risparmi di una vita? L'importante è aiutare le banche, perché poi vi ritornerà utile e sappiamo come. E per la casta? Oh, per la casta i soldi ci sono e ci devono essere sempre. In questi anni avete costruito un mondo a parte, fatto di privilegi che i comuni cittadini neanche immaginano e neanche conoscono tutti. Ma in questa XVII legislatura qualcosa è cambiato: siamo entrati noi in Parlamento, noi, quelli che voi chiamate populisti, antipolitica e una serie infinita di altri appellativi. Ci additate con fare sprezzante per cercare di fare presa sull'opinione pubblica e nascondere così il vergognoso piccolo regno che vi siete creati qui. Siamo riusciti in questa legislatura, nonostante fossimo e siamo all'opposizione, a mettervi nella condizione, anzi a obbligarvi a parlare e a effettuare azioni concrete per un taglio reale dei costi della politica. E abbiamo iniziato a smussare alcuni dei privilegi che vi stanno tanto a cuore. La scorsa settimana, dopo quasi un'intera legislatura - quattro anni e quattro mesi, per l'esattezza - e grazie alle pressioni del Movimento 5 Stelle, è stata approvata in prima lettura dalla Camera una legge che abolisce i vitalizi e prevede il ricalcolo pensionistico per i parlamentari su base contributiva. Il provvedimento adesso è arrivato qui in Senato e abbiamo visto proprio oggi come la cosa vi abbia reso felici e come avete reagito, visto che avete bocciato la richiesta di dichiarazione di urgenza del provvedimento, preferendo rinviare a settembre per cercare di allontanare quanto più possibile da voi questo fausto evento. Ma, in merito a questo, vorrei specificare che quanto detto stamani dal presidente Zanda ha davvero del tragicomico. Egli infatti ha chiesto perché avessimo presentato proprio ora, a poche ore dalla sospensione dei nostri lavori, una richiesta di dichiarazione di urgenza. La risposta è semplice: ora è stato incardinato il provvedimento in Commissione. Vorrei ricordare al senatore Zanda che sono loro gli esperti di queste furbate, non noi. Zanda si è forse dimenticato che avete voluto e costretto l'Aula a incardinare la legge elettorale il 20 dicembre 2014 alle ore 7,39 del mattino, prima della pausa di Natale? Legge, fra l'altro, dichiarata incostituzionale, come quasi tutte quelle volute da questa maggioranza. Comunque rassegnatevi: settembre è vicino. Ma non è l'unica cosa a cui abbiamo posto la parola fine. Mi riferisco - ad esempio - agli affitti d'oro. Vi ricordate? Spendevamo 30 milioni di euro per questi e noi li abbiamo fatti saltare. Addirittura era prevista un'assicurazione per i parlamentari per le punture di insetti e per questo venivano spesi 350.000 euro alla Camera dei deputati. Ma come? Agli italiani per l'assistenza sanitaria volete far pagare ormai tutto, anche a chi ha la pensione minima, e per voi avevate previsto addirittura un'assicurazione per le punture di insetti? Ma vi rendete conto dell'assurdità di questa cosa? Viene vergogna anche solo a riportarla a voce. E voi un po' di vergogna quando la volete mostrare? Non parliamo poi delle auto blu e dei tanti altri privilegi che vi siete creati *ad hoc*. Ma c'è tanto ancora da fare, perché questo Parlamento è un pozzo senza fondo, fatto di privilegi. E allora veniamo nello specifico al Senato, e mi rivolgo ai cittadini che ci seguono da casa. Sapete che nel bilancio del Senato - ad esempio - c'è una voce di spesa, la 01.17.01 (Servizi di mobilità), per ben 400.000 euro annui, destinati al rimborso dei biglietti aerei e ferroviari dei senatori cessati dal mandato da non più di dieci anni? Sì, avete sentito bene: i privilegi rimangono anche quando non sei più un parlamentare in carica. Come Movimento 5 Stelle crediamo che questo sia inaccettabile e incomprensibile. Perché mai lo Stato e i cittadini devono farsi carico di spese di viaggio di una persona che non svolge più una funzione pubblica, ma anzi è cessata dalla carica? Non vi sono forse bastati i soldi che già avete percepito durante il mandato? Ci potete chiamare come volete, ma intanto - e gli italiani lo sanno - siamo gli unici - e ripeto: gli unici - ad aver rinunciato a 42 milioni di rimborsi elettorali, mentre voi ve li siete intascati tutti. luogo, siamo gli unici a esserci dimezzati gli stipendi e a restituire anche le diarie in eccedenza, mettendoli al servizio dei cittadini attraverso il microcredito. Grazie ai 22 milioni di euro raccolti - e parlo solo delle restituzioni di noi parlamentari parlamentari - sono nate oltre 6.100 nuove aziende, per circa 14.000 nuovi posti di lavoro. Vi sembra poco? Forse. Ma la domanda è: voi che cosa avete fatto? Di sicuro queste sono cose che vogliamo diventino la regola e lo diventeranno di sicuro quando saremo noi al Governo. Quindi preparatevi. Concludo, signor Presidente. con questo ordine del giorno noi proseguiamo nella nostra azione di azzeramento dei privilegi della casta, che non hanno alcun fondamento e ragione di esistere. Per tale motivo, chiediamo che il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori si impegnino a eliminare dal bilancio del Senato, a partire dalla XVIII legislatura, tutte le spese relative al rimborso dei biglietti aerei e ferroviari dei senatori cessati dal mandato. Quindi, colleghi, mettetevi una mano sulla coscienza e cercate di essere ragionevoli.

dell'economia. Essa si rende necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini all'istituzione parlamentare, in armonia con l'andamento economico per nulla esaltante del Paese. Secondo i dati ufficiali dell'ISTAT, a giugno la disoccupazione si attesta all'11,1 per cento: una percentuale che, pur essendo leggermente in calo, è ancora elevata

nel 2016: sono 1.619.000 le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta. queste cifre ci sono persone, famiglie, soprattutto quelle con minori, che quotidianamente, tra mille difficoltà, devono pensare ad arrivare a fine mese, senza peraltro neanche riuscirci in molti casi. L'articolo 69 della Costituzione dispone che i membri del Parlamento ricevano un'indennità stabilita dalla legge. Ciononostante, attraverso l'adozione di regolamenti interni delle Camere, si è istituito altresì un regime speciale di tipo previdenziale per i deputati e i senatori. In particolare, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 289 del 1994 ha precisato come l'evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa particolare forma di previdenza ha condotto anche a configurare l'assegno vitalizio come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito in parte aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private. Inoltre, - precisa la Corte - tra l'assegno vitalizio e il trattamento pensionistico non sussiste un'identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che, a differenza della pensione ordinaria, l'assegno vitalizio viene a collegarsi a un'indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto nella disciplina costituzionale e ordinaria connotazioni distinte da quelle della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego. In altri termini, il mandato parlamentare, non configurandosi come un impiego pubblico, bensì come l'esplicazione di una missione pubblica in rappresentanza della Nazione, non può e non deve essere assistito assistito da un regime pensionistico assistenziale in aggiunta alla costituzionalmente necessaria indennità. per quanto concerne il capitolo riferito al trattamento dei senatori cessati dal mandato, il bilancio di previsione prevede una spesa di 83 milioni di euro per l'anno 2017, perfettamente invariata rispetto all'anno precedente. Di fronte a queste cifre, e soprattutto rispetto all'attuale crisi della quale ho parlato prima, è del tutto opportuno che anche i senatori contribuiscano al contenimento della spesa del Senato. È vero che alla Camera dei deputati la scorsa settimana è stata approvata la proposta di legge che ricalcola i vitalizi, ma il fatto che oggi abbiamo respinto l'esigenza di doverla esaminare con urgenza, e poiché la legislatura volge al suo termine ed è molto difficile che la proposta diventi legge a tutti gli effetti, è necessario, al contrario, un contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato che la Corte costituzionale ha peraltro riconosciuto la Corte costituzionale ha peraltro riconosciuto come compatibile con il dettato costituzionale. Quindi, tale contributo potrebbe essere attivato con una delibera del Consiglio di Presidenza, e in particolare del Collegio dei senatori assoggettando gli assegni vitalizi erogati a favore dei senatori e dei loro familiari ad un contributo di perequazione pari al 20 per cento per importi lordi fino a 90.000

La pubblicità dei lavori parlamentari rappresenta un principio costituzionale di fondamentale importanza ed è sempre più ineludibile la necessità di trasformare queste istituzioni in veri e propri palazzi di vetro. In questa direzione il Senato della Repubblica è impegnato nel garantire la pubblicità dei lavori. Ad oggi, tuttavia, non è ancora stata prevista la pubblicità sul sito *web* dell'attività del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Questori, il cui contenuto, pertanto, rimane inaccessibile ai cittadini. Nel corso dell'esame del bilancio interno del Senato dell'anno 2016 è stato approvato un ordine del giorno del giorno volto a impegnare, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a studiare i criteri per la pubblicazione di di interesse generale adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Collegio dei Questori nel corso della legislatura. Con l'ordine del giorno G47 si vuole pertanto impegnare il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori, ognuno per le proprie rispettive competenze,

disincentivi di carattere regolamentare sui quali la Giunta per il Regolamento sta già lavorando, è di provare a mettere in campo anche disincentivi di carattere economico. Il disincentivo di carattere economico proposto, nei limiti di questo ordine del giorno e delle competenze del Consiglio di Presidenza, è quello di non computare nel calcolo del contributo versato al Gruppo parlamentare i senatori eventualmente aggiunti perché si sono spostati da un Gruppo all'altro, così da disincentivare le

di provenienza, perché molto spesso questa situazione fa sì che Gruppi che hanno preso impegni di bilancio anche con i dipendenti, quindi con le risorse umane, si trovano ad avere una carenza e non possono più

per la precisione, esso verte sulla richiesta di centralizzazione della contrattualizzazione dei collaboratori parlamentari. In soldoni, ciò significa fare in modo che l'istituzione Senato gestisca internamente l'assunzione di tutti i collaboratori parlamentari, esattamente come succede per i collaboratori del Consiglio di Presidenza, del Collegio È una cosa che avrebbe notevoli impatti positivi. Abbiamo ascoltato prima, sia dal Presidente della 5ª Commissione che dal Collegio dei Questori, tutta una serie di numeri sui

si avrebbe una rivalutazione di queste figure professionali. La stessa cosa succede già nel Parlamento europeo e nella stragrande maggioranza dei Consigli regionali.

altri senatori e altre senatrici hanno evidenziato il forte ritardo nella presentazione, non tanto del rendiconto, quanto del bilancio preventivo,

Non ne discuto la legittimità, perché c'è anche un decreto del Presidente del Senato che autorizza l'esercizio provvisorio, ma ritengo che non sia opportuno e non sia comunque elegante accumulare un ritardo così vistoso, tenuto conto che agiamo con uno strumento contabile di cassa. È vero che la contabilità della pubblica amministrazione è sottoposta - dico io, purtroppo ad altre regole rispetto a quelle dei privati, ma un'azienda di servizi industriali che presentasse un*budget* a oltre metà dell'esercizio sarebbe sicuramente punita da qualcuno: dall'azionista, dall'assemblea dei soci, dai C'è, però, un'osservazione di merito che mi interessa maggiormente esprimere e per cui ho chiesto la parola questa sera. Intanto, vorrei ringraziare il Collegio dei Questori e, ovviamente, la Presidenza per il lavoro che hanno svolto in questi quattro anni e mezzo; ringraziarli per la qualità del lavoro svolto e per il modo con cui hanno operato, dalle scelte economiche, a quelle logistiche, agli interventi in Aula, in una legislatura non facile, in cui si sono scomposti e costituiti nuovi Gruppi.

obiettivo particolarmente avvertito in questa stagione storica, cioè il contenimento dei costi. Nella relazione di accompagnamento si evidenzia questa minore spesa, che dal 2013 a oggi si aggira intorno ai 190 milioni La spesa del Senato, dunque, segue da anni un *trend* decrescente. Signor Presidente, probabilmente c'era del grasso. Si sono realizzate delle economie di scala, su versanti non produttivi. Si sono realizzate economie razionalizzando la struttura organizzativa, però la domanda - ecco il motivo del mio intervento che io pongo all'Assemblea e ovviamente a chi gestirà i bilanci futuri è la seguente: c'è un punto limite di caduta?

Certo, nelle istituzioni pubbliche contano anche l'immagine, i segnali e gli esempi, ma un'azienda che fa scarsa manutenzione ai propri impianti, non fa investimenti e taglia sul personale, non attuando il *turnover*, conquista o perde o perde il mercato di riferimento? Non ho fatto a caso l'esempio di un'azienda e dei suoi centri di costo. Ci sono parti consistenti di Palazzo Madama - mi fermo qui

Nell'area relativa al personale si registrano consistenti risparmi, che sono stati portati, non dico come esempio, ma come fatto virtuoso. Noi tutti riconosciamo al personale di quest'Istituzione professionalità, impegno e dedizione, ma se scaviamo in profondità ci accorgiamo che siamo al limite, forse anche oltre, in alcuni servizi di Assemblea e di Commissione, nonché nei servizi amministrativi. Il blocco del *turnover* altera anche la qualità del prodotto. Qui si fanno leggi, non si producono succhi di frutta. Per rimanere sempre a questo esempio dei succhi di frutta, il declino di un'impresa si nota subito, perché sul mercato quel prodotto non si vende più.

Signor Presidente, grazie della disponibilità e del tempo ulteriore

le parti e gli operatori hanno accesso e disponibilità, oltre che alle norme da applicare, anche ai precedenti, alla giurisprudenza

di rendere pubblici i precedenti parlamentari riferiti agli articoli del Regolamento del Senato e alle loro diverse interpretazioni, sulla base delle precedenti prassi applicative. È infatti assolutamente noto che nell'ambito dei lavori parlamentari il valore della prassi e del precedente assume una importanza primaria e prioritaria, che talvolta giunge a svuotare la norma regolamentare scritta.

Tale potere - peraltro assolutamente legittimo - gli deriva infatti dal fatto di disporre di tutti i precedenti e delle prassi con assoluta immediatezza. La trasparenza deve rappresentare un valore fondamentale della nostra Assemblea e del nostro Regolamento: la sua conoscenza e la sua l'applicabilità deve, dunque, essere accessibile a tutti. Questo lo dico tanto più alla luce della probabile nuova giurisprudenza che magari si svilupperà quando, auspicabilmente, la Giunta per il Regolamento licenzierà un nuovo testo del Regolamento del Senato con delle modifiche e quindi sarà ancora più importante disporre fin da ora

i numeri di bilancio che il Collegio dei Questori ha presentato in realtà non fanno altro che confermare, sia nel consuntivo che nel preventivo, il lavoro che il Collegio dei Questori ed il Consiglio di Presidenza nella sua interezza hanno fatto in questi anni, orientato alla razionalizzazione delle spese, provando ad eliminare sprechi e a ridurre i costi generali senza farne venire meno la funzionalità. I numeri ovviamente sono positivi, ma dovremmo provare a leggere i contenuti che sottendono a questi dati, anche partendo dal presupposto che ci troviamo in una fase totalmente diversa da quella precedente. Lo scorso 4 dicembre, come hanno ricordato altri colleghi, i cittadini italiani hanno bocciato la riforma costituzionale promossa dal Governo Renzi, che prevedeva anche l'abolizione - in realtà una falsata narrazione - di questa Istituzione. Si è raccontato che con l'abolizione del Senato il nostro Paese avrebbe avuto risparmi enormi ed avremmo risolto tutti i problemi. Per fortuna, i cittadini hanno respinto il *referendum* e ancora una volta - dico per fortuna - si sta proseguendo nell'azione di razionalizzazione delle risorse pubbliche per evitare soprattutto gli sprechi. A noi, dunque, spetta, attraverso i numeri, il compito di consolidare un'istituzione democratica, fondamentale per questo Paese, che nel corso della sua lunga storia, quando gli è stato possibile e persino in questa legislatura nonostante il continuo ricorso alla fiducia, ha svolto un lavoro legislativo importante. Un lavoro che non nasce solo dall'impegno di noi senatori e delle forze politiche, ma anche dall'impegno delle tante persone, dei tanti lavoratori e lavoratrici che sono impegnati con passione, professionalità e competenza, e spesso oltre le loro funzioni. Siamo all'ultimo bilancio di questa legislatura e non possiamo perdere l'opportunità di ringraziare tutti e tutte, ma abbiamo anche il dovere di prendere degli impegni. Pochi, non tanti, ma impegni veri. Ed allora non possiamo non riconoscere che la cura dimagrante del personale, in parte dovuta ai pensionamenti, che ha consentito in dieci anni di passare da 1.098 dipendenti a 651, è stata accompagnata anche da forme di esternalizzazione di servizi importanti, dai servizi tecnici tecnici delle votazioni, ai servizi di portineria, ai servizi di pulizie, bar e mensa (e sicuramente ne dimentico molti altri). Non solo non ci sono dati che confermano che abbiamo risparmiato attraverso le esternalizzazioni - e vorrei che non fosse solo una valutazione economica, ma anche una valutazione tra costi e benefici - ma di sicuro abbiamo contribuito ad accrescere il lavoro precario ed insicuro. Il Senato della Repubblica non può essere il luogo dove i processi di esternalizzazione rischiano di diventare prassi o dove persiste il precariato. Per questo motivo abbiamo presentato un ordine

scadenza della legislatura. Questi impegni consentirebbero di sanare un *vulnus* che si trascina da anni e di cui, addirittura, si sono perse le origini. Per questo il Senato ha necessità di proseguire il suo cammino su basi solide e con il sostegno di tutte le professionalità presenti,

Zanda. Il presidente Zanda ha finalmente riconosciuto il ruolo di questa Camera, che non deve essere quello di un semplice passacarte. In realtà, io mi ero un po' confusa in questi quattro anni e mezzo di mandato perché di fatto, molto spesso, abbiamo fatto proprio i passacarte del Governo, che fosse quello di Renzi, quello di Letta o quello di Gentiloni Silveri. Noi non abbiamo fatto altro che ratificare.

E questo atto di imperio è arrivato addirittura dalla banca stessa, e neanche dal Governo. Quindi, sentir riconoscere finalmente un po' di dignità a questa Camera ci ha fatto molto piacere. È poi anche giusto che si possano approfondire il provvedimenti e che i senatori e le senatrici possano avere il tempo opportuno per approfondire tutte le leggi e tutti i provvedimenti che questa Camera adotta. Io mi auguro che così sarà anche, per esempio, per il rendiconto dello Stato, che è stato incardinato oggi in Commissione. Abbiamo un mese di tempo, quello delle vacanze. Peccato che il rendiconto dello Stato sia formato da diversi tomi e da migliaia di pagine che dovrebbero essere puntualmente analizzate dai senatori, prima di essere approvate o respinte. Invece la legge sui vitalizi consta di pochi articoli e pochi concetti, però per quelli si è richiesto un tempo infinitamente più lungo; ma va bene così. L'ordine del giorno G60, per cui chiedo l'approvazione, impegna a pubblicare l'elenco dei soggetti che nel corso di questa legislatura hanno beneficiato di elargizioni e dei senatori che ne hanno disposto l'erogazione. Questi contributi e sussidi ammontano esattamente a 1.262.500 euro. Ebbene, è strano che, di tanta puntualità, correttezza e rispetto delle istituzioni che viene dai banchi di quest'Aula nel momento in cui si richiede l'abolizione dei vitalizi, si dia più di un milione di euro appannaggio ‑ così si dice ‑ di alcuni senatori, somme che poi questi dispensano e regalano a chissà chi, senza che i colleghi ne abbiano contezza, ma, cosa ancor più grave, senza che i cittadini sappiano a chi vanno questi soldi. Dobbiamo infatti puntualizzare che di oltre un milione di euro non viene mica dalle casse del Partito Democratico, di Forza Italia o di tutte quelle forze che oggi hanno impedito la calendarizzazione d'urgenza dell'abolizione dei vitalizi, ma viene esattamente dalle tasche dei cittadini. Quindi, sono certa che non ci sarà nessuna opposizione in merito all'approvazione

che tutti abbiano fornito un importante contributo all'attività che ci troviamo a gestire durante l'anno. Naturalmente mi associo - e non mi dilungo perché lo ha già fatto autorevolmente il questore De Poli - anche ai ringraziamenti a tutti coloro che contribuiscono al buon andamento del Senato.

e l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito della sfera di autonoma determinazione ad essi riservata dal Regolamento del Senato e nell'ambito della recente costituzione del ruolo unico,

la formazione continua viene fatta regolarmente e tale formulazione potrebbe non essere consona.

seguente: «a valutare l'opportunità di procedere, anche alla luce delle integrazioni funzionali con l'Amministrazione della Camera, definite con i protocolli sottoposti alla deliberazione ufficiale del Consiglio di Presidenza nella riunione del 10 maggio 2017, a ulteriori interventi di riorganizzazione funzionale o organizzativa che risultino idonei ad accrescere l'efficienza e l'economicità delle attività di supporto svolte dall'Amministrazione». Anche in questo caso la riformulazione

del giorno G6 si chiede di rideterminare l'indennità parlamentare e altre indennità accessorie. Il parere è contrario. Già c'è stata una riduzione nel corso degli anni del 30

nel passato; riteniamo che sia logico che ne resti traccia per un principio normale che c'è in qualunque amministrazione per cui a incarichi

G10 chiedono sostanzialmente una rendicontazione generale. Ricordo che recentemente è stata introdotta la rendicontazione di una parte importante di questi rimborsi inoltre, che non c'è alcun Parlamento dell'Unione europea che preveda una rendicontazione di questo genere. Ci sono, invece, cifre forfetarie,

relativa per il personale, ma con somme molto più alte delle nostre: il Parlamento europeo, al posto dei nostri 4.000 euro che comprendono anche altri tipi di spese, arriva a 24.000 euro; il Bundestag tedesco prevede 19.000 euro;

G11 il parere è contrario perché è chiaro che nell'esercizio del mandato del parlamentare c'è la collaborazione con i soggetti politici, con i partiti e con con i movimenti nell'ambito dei quali si esplica - credo non ci siano eccezioni in questa Aula - la maggior parte del lavoro parlamentare. Per cui, è perfettamente normale che il modo in cui i parlamentari contribuiscono, spesso in maniera decisiva alla vita dei soggetti politici che sono riconosciuti - lo ricordo - dalla Costituzione, sia una delle voci più specifiche per le quali sono erogati i fondi per il rimborso del mandato. Pertanto, il parere è contrario.

per via dell'evoluzione dei prezzi nel mercato delle telecomunicazioni, ma è anche vero che l'altra parte di spese generali, rappresentata dai viaggi di spostamento all'interno del collegio o dell'intero Paese (dal momento che ai sensi della Costituzione rappresentiamo l'intero Paese) è invece particolarmente aumentata e in particolare sono salite alle stelle le tariffe di parcheggio presso gli aeroporti. È dunque perfettamente normale che quella

a seguito di una delibera del 2009, è stata ridotta dell'80 per cento per via della riduzione degli importi, cioè per il fatto di aver legato questo tipo di rimborsi non al numero di viaggi, ma alla spesa effettivamente sostenuta, ed è limitata nel tempo. Pertanto, che un ex senatore possa vedersi rimborsate le spese per venir a dare il suo contributo a partecipare a convegni o ad attività

studiare modalità per regolamentare regali e utilità ricevute in virtù della carica ricoperta.

perché l'assegno di fine mandato non è nel bilancio del Senato, ma in un fondo a parte. Queste sono somme accantonate rispetto all'indennità che percepiscono i senatori, quindi sono di loro proprietà esattamente come gli esattamente come gli analoghi trattamenti che ci sono per i lavoratori dipendenti. Faccio presente che si tratta di un istituto presente anche in Parlamenti di Paesi nei quali non c'è il trattamento di fine rapporto per i lavoratori, perché ha una valenza particolare.

siano inammissibili perché rientrano in ambiti che già sentenze della Corte costituzionale hanno stabilito che non possono essere affrontati o, quanto meno, non possono essere affrontati in questo modo. come abbiamo visto questa mattina, la questione viene ampiamente affrontata da un disegno di legge che è all'esame proprio del Senato. Pertanto ritengo che tali ordini del giorno, in analogia con quanto è già stato fatto negli anni scorsi sia al Senato, sia nell'altro ramo del Parlamento, siano inammissibili. Per quanto riguarda

G27 propone di tornare ad intervenire sulle pensioni dei parlamentari colpiti da condanne per alcuni reati. Si tratta - come dice l'ordine del giorno stesso - di una decisione del Consiglio di Presidenza molto recente (7 maggio 2015), che è avvenuta dopo un ampio dibattito e uno studio approfondito. Non ritengo che sia opportuno reintervenire sullo stesso argomento, visto che è già stato oggetto di recente dibattito; esprimo pertanto un parere contrario. G28, l'elenco dei percettori delle pensioni parlamentari è già disponibile sul sito del Senato. Per quanto riguarda gli importi, del senatore Santangelo)*. Sappiamo che tutti i giornali lo fanno, ma lo fanno sulla base di un semplice calcolo: conoscendo quali sono le norme, si fa presto a calcolare quanto percepisce chi ha fatto uno, due, tre mandati e così via.

fin dall'inizio della legislatura, in modo organico e definitivo. Il presidente Grasso rinuncia a usare una parte molto importante di queste dotazioni. di queste dotazioni. Ritengo peraltro che non sia logico che il Presidente del Senato italiano, che è anche vice Presidente della Repubblica a tutti gli effetti, abbia una dotazione inferiore a quella di un qualunque senatore degli Stati Uniti. Per cui esprimo parere contrario

somme di voci del bilancio già ridotte del 30 per cento per decisione del Consiglio di Presidenza. In particolare, le indennità per gli ex Presidenti del Senato sono state ridotte nell'entità e nella durata

in tutta questa legislatura si è sempre registrato un lieve avanzo di questo fondo, che è alimentato dai versamenti dei senatori. Il parere è invece contrario sulla prima parte dell'ordine del giorno G32,

del giorno G35, G36 e G37 si riferiscono in modo diversi alla questione dei senatori

quanto per tutte quelle risorse che vengono versate come contributo ai Gruppi, ma che stanno in capo all'attività di ciascun singolo senatore.

nel nuovo Gruppo, e voi intervenite cambiandolo proporzionalmente anche durante l'anno, quindi a seconda di quanto tempo il senatore è stato in un Gruppo o in un altro. Siccome il Regolamento non dice nulla in tal senso, si potrebbe anche intervenire esclusivamente con una deliberazione del Consiglio di Presidenza e non necessariamente per via regolamentare. Magari si potesse intervenire anche per Regolamento! Quello ce lo augureremmo, ma in altre sedi. Qui è comunque un'indicazione, e per questo non lo ritiriamo.

giorno G39, G40 e G41, in modi diversi affrontano il problema di varie forme di precariato.

perché contraddicono il principio per cui al Senato si entra per concorso, ben comprendendo le tematiche sollevate. Faccio anche notare che ci sono tuttora delle tutele per alcuni di questi casi, in particolare il famoso personale *ex* delibera n. 58 del 1993. Purtroppo, non si può andare oltre per via del principio del concorso che peraltro riguarda il Senato, ma è anche un principio generale della pubblica amministrazione.

Nell'ordine del giorno G43 si afferma che attualmente gli incarichi vengono attribuiti in modo generalizzato senza rispondere sostanzialmente a criteri di buona amministrazione, per cui il parere contrario è insito nella formulazione stessa del testo.

tale sistema, che già viene applicato, va integrato insieme alla Camera, alla luce delle decisioni recentemente intervenute. Esprimo parere contrario sull'ordine contrario all'attuale ordinamento del Senato, che prevede una figura di vertice di riferimento. Esprimo parere contrario

per la verità, assai di rado - in altri rami della pubblica amministrazione, in quanto sono necessarie in alcuni casi delle specializzazioni e la continuità dell'amministrazione necessita, dato anche il numero molto ridotto del personale, di intervenire in questo senso.

per la pubblicazione di delibere del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Questori di interesse generale». È una cosa da attuare perché ci sia un puntuale rendicontazione e consultabilità di queste decisioni, che naturalmente devono salvaguardare la *privacy*. Non può evidentemente essere accolta la prima parte dell'ordine del giorno G47, che prevede addirittura la pubblicazione di resoconti integrali. Ricordo che ci sono organismi, come il Consiglio dei Ministri, le Giunte regionali, comunali e quant'altro, che non prevedono questa resocontazione, per la natura assai simile a quella del Consiglio di Presidenza. Mentre la pubblicazione

per cui noi, tanto più come Questori, non possiamo certamente prendere l'impegno di pubblicare qualcosa che non c'è. E se ci fosse, dovrebbe essere regolamentata, perché diventa una sorta di

del giorno G53 è accolto come raccomandazione per le parti compatibili con l'ordinamento del Senato. perché gran parte delle norme cui fa riferimento il presente ordine del giorno non sono usate dal Senato: non ci sono dirigenti esterni nominati, come invece è previsto

G54 elenca voci sulle quali si spende meno della metà degli stanziamenti che ci sono, che però, per occasioni particolari, potrebbero formulare necessità dell'uso, pertanto esprimo parere contrario: si tratta di un bilancio, non della

alla complessiva dotazione.

G56 propongo una riformulazione: «a valutare ulteriori interventi, dopo quelli già realizzati, di razionalizzazione nella programmazione degli eventi presso le sale del Senato».

tenendo presente che alcune di queste voci sono proprio a zero, come il famoso contributo al circolo di Palazzo Madama, parere è contrario: si tratta di voci già ridotte o comunque utilizzate attualmente in maniera estremamente limitata. G63 e G64 il parere è favorevole: è una cosa che già si fa ed è giusto continuare in questa direzione.

G66 è accolto come raccomandazione, per verificare la fattibilità materiale di questa iniziativa. Sull'ordine G68: raccogliamo anche la particolare sollecitazione che vi è stata su questo punto, che rappresenta davvero uno degli aspetti fondamentali della vita del Senato, ossia il controllo del complesso

Alla luce dei pareri espressi, gli ordini del giorno G18, G19, G16, G17, G20, G21, G22, G23, G24, G25, G40 G40 e G41 sono dichiarati inammissibili. Gli ordini del giorno G50 e G51 sono dichiarati improponibili per estraneità all'oggetto della discussione. Essendo stati

ad eliminare dalle voci di spesa ammissibili ai fini del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, le somme versate dai Senatori ai soggetti politici sia a titolo di erogazione liberale, sia quale corrispettivo o rimborso della fornitura di servizi e prestazioni ricevute. Non diciamo che queste somme non devono essere date, ma che i 2.090 euro rendicontati non devono essere contabilizzati. Vi dico anche perché. Se rendiconto 2.090 euro di contributo al partito, al partito, non ho bisogno di rendicontare i rimanenti. Quindi, se utilizzo dei sistemi anche un po' *borderline* per pagare i collaboratori o fare dei contratti, non c'è la possibilità di fare le verifiche.

Aggiungo un ulteriore particolare, che forse molti dimenticano. Queste erogazioni liberali vengono poi inserite nel modello unico per avere l'ulteriore detrazione del 19 per cento Sì, perché non c'è alcun motivo per non farlo, perché la legge lo prevede. Se io ho versato dei contributi liberali al partito, questi sono oggetto di deduzione nel modello unico. Quindi, non solo si prendono 4.180 euro, ma anche la detrazione del 19 per cento dalle tasse nel modello unico. Signor Presidente, mi creda, è così è così e sfido chiunque a vedere le dichiarazioni delle deduzioni e detrazioni. Le dichiarazioni dei redditi sono pubbliche sul sito. Andate a controllare e verificare se non è così.

la trasparenza non è mai negativa. È sempre una buona cosa, anche per le spese sanitarie, magari, perché so che ci sono alcuni parlamentari, anche del mio ex partito, che contano due

ma di azzerare qualsiasi attribuzione spettante agli ex Presidenti del Senato. Mi dispiace per l'attuale Presidente del Senato, che magari potrebbe

mentre l'ordine del giorno della senatrice Comaroli faceva giustamente una distinzione tra quelli che si sono movimentati all'interno del Senato per propria volontà e quelli che, invece, lo hanno fatto in modo non volontario, io, ricordando al senatore Crimi che, se voleva evitare di perdere tutto quel denaro che dice aver perso il suo Gruppo, bastava che non buttasse fuori qualche decina di persone. Semmai, avrei votato a favore se fosse stato previsto un indennizzo per chi è stato buttato fuori. Quindi, il mio voto sarebbe stato contrario.

PLI))*. Signor Presidente, vorrei ringraziare innanzitutto il Consiglio di Presidenza e i senatori Questori per la qualità del bilancio che hanno presentato oggi a quest'Assemblea: è evidente che su un tale complesso atto essi hanno lavorato con costanza, capacità e serietà, orientando il documento alla contrazione costante della spesa. Spiccano, sulle altre, alcune cifre che in questo senso sono determinanti e offrono una lettura chiara e precisa: 188 sono i milioni di euro risparmiati, suddivisi tra i 108 milioni di minori risorse sollecitate allo Stato e gli 80 milioni di ulteriori risparmi che allo Stato verranno restituiti. Il Senato ha tagliato la spesa complessiva agendo su più fronti, attuando misure di contenimento della spesa in ogni ambito, dalle uscite per i senatori a quelle per il personale, a quelle per il funzionamento della macchina amministrativa. Per esaminare soltanto il primo dei capitoli appena citati, quello che ci riguarda più da vicino, va osservato con favore che il rapporto tra la spesa per le indennità dei senatori e il bilancio del Senato è passato dal 2001 al 2017 dal 19 per e quindi risulta praticamente dimezzato. E siccome le cifre non sono opinabili, 37,2 milioni di risparmi che troviamo nel bilancio che stiamo esaminando sono un fatto concreto di cui dobbiamo tenere conto nella nostra valutazione. Così come sento di sottolineare un altro dato tra quelli che ci sono stati illustrati poco fa: il rapporto tra la spesa del Senato e il bilancio dello Stato oggi continua a scendere (dallo 0,083 del 2007 allo 0,059 del 2016; in pratica, per ogni mille euro spesi dallo Stato, Palazzo Madama spende 59 centesimi). Naturalmente, come accade in ogni organizzazione, sia privata che pubblica, ciò che rileva davvero e finisce per essere la variabile dirimente, è quanto la spesa sia giustificata dalla produttività. Al di là della retorica, colleghi, mi sento di affermare, senza tema di smentita, che su questo punto la valutazione la dovranno fare in nostra vece i cittadini Dico questo perché voglio farmi portatore di un auspicio, che condivido con tutti i componenti del mio Gruppo, Federazione della Libertà. Vorremmo fortemente che dal Senato giungesse un messaggio positivo per tutti gli italiani, fuori da questo prestigioso Palazzo, che proprio gli italiani hanno proprio gli italiani hanno voluto - e il segnale è stato forte e chiaro - che proseguisse il suo lavoro e conservasse il suo fondamentale ruolo istituzionale. Dunque la strategia seguita, di deciso contenimento della spesa, ha raccolto un messaggio che proprio dalla cittadinanza arrivava, anch'esso forte e chiaro. Questa Camera lancia così un messaggio distensivo e contribuisce a costruire un ponte che

a quanti vivono in condizione di povertà - è indispensabile che le istituzioni facciano la propria parte sul fronte del contenimento della spesa e sul consequenziale migliore impiego delle risorse. È evidente che questa sfida il Senato la sta già cercando di vincere e con numeri importanti, che cristallizzano il fatto che una istituzione che punta sull'innovazione e sulla modernizzazione, proprio come un'azienda diligente, può migliorare i processi produttivi e ottimizzare le risorse. Da queste semplici considerazioni ne scaturisce un'altra: noi qui, più di chiunque altro, abbiamo il dovere di essere sempre più trasparenti, di aprire il Palazzo ai cittadini. Il "nuovo" Palazzo Madama, il Senato nella sua immagine nuova, quella che noi tutti stiamo impegnandoci a dare, ha l'ambizione di diventare un'istituzione sempre più leggera, sempre più dinamica, capace di veloci scatti in avanti, in piena sintonia con il Paese che rappresenta. Signora Presidente, colleghi senatori Questori, è inoltre necessario che ognuno di noi - e il Senato nella sua collettività - si impegni sempre più a garantire la massima trasparenza sulle entrate e le uscite, a dimostrazione che l'utilizzo delle risorse avviene nel modo più oculato e corretto possibile. Il medesimo sforzo lo si deve certamente richiedere anche nella gestione delle risorse all'interno dei Gruppi e dei servizi - chiamiamoli così - *pro* quota di cui i singoli senatori possono disporre per i propri uffici, magari proprio evitando quegli inutili doppioni di cui si è parlato anche durante il dibattito. In particolare, bisogna fare in modo che la democrazia alberghi il più possibile anche all'interno dei Gruppi parlamentari e che non vi sia, dunque, la possibilità di discriminare eventuali posizioni dissidenti. In altri termini, a me pare che la legge ferrea delle oligarchie, troppe volte, viga ancora in alcuni Gruppi e ancor di più nei partiti. Ma questo, colleghi, mi rendo conto, è un capitolo che apriremo e approfondiremo nelle sedi opportune e in particolare in sede di discussione e aggiornamento del Regolamento del Senato, che risulta sempre più urgente per snellire e rendere più efficace questa Camera. Questa dell'esame del bilancio di previsione 2017, insieme al rendiconto del 2016, è una occasione anche per tirare le somme su cinque anni di legislatura, anni durante i quali, giorno dopo giorno, abbiamo assistito e partecipato a importanti cambiamenti, sovente su piccoli aspetti che non incrementano i numeri, ma che conquistano la loro importanza nel momento in cui avvicinano gradualmente gli italiani al lavoro del Senato. Vale qui la pena ricordare i notevoli passi avanti sul fronte della fruibilità delle sedute dell'Aula e delle Commissioni. Grazie alle potenzialità, alcune ancora da dispiegarsi, del *web*, il Palazzo è a portata di clic e la partecipazione democratica ne è esponenzialmente favorita e quanto sia sempre forte il desiderio di partecipazione è dimostrato dai 23 milioni di visualizzazioni in questa legislatura, sempre più trasparente e accessibile a tutti. In ultimo, vengo a un capitolo che ha modificato anche le nostre abitudini, ha velocizzato il lavoro di tutti e ha contribuito alla diminuzione sensibile dell'impatto ambientale: la dematerializzazione degli atti parlamentari, che ha ridotto del 75 per e aperto la strada all'accesso a tutti gli atti in formato elettronico, facilmente riproducibili e massimamente condivisibili. Si tratta di un piccolo cambiamento, che è segno dei tempi. Con l'auspicio che il lavoro svolto - e mi avvio alla conclusione - possa continuare con la stessa determinazione, energia e incisività nella prossima legislatura, confidiamo, cari colleghi, nella condivisione e nella collaborazione da parte di tutte le forze politiche rappresentate in quest'Aula. Intanto, a nome di tutti i componenti, annuncio con piacere il voto favorevole a nome del Gruppo Federazione della Libertà al rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2016 e al progetto di bilancio interno per l'anno finanziario 2017. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI))*.

come i senatori siano al centro molte volte di critiche, cui dobbiamo stare attenti,

termine. Per tutte queste motivazioni, facendo riferimento anche alla relazione del senatore Tonini su quelle che una volta erano le spese

non rilevare un miglioramento, ovvero un contenimento dei costi; rimangono però alcuni aspetti di carattere tendenziale che credo vadano messi in evidenza. Intanto, su un totale di 492 milioni di euro di spesa, nel 2016 le spese di funzionamento - come ci ha ricordato il presidente Tonini

Ciò è molto evidente nel dato relativo ai trattamenti pensionistici del personale, che passano dai 119,9 milioni del 2014 ai 142,323 del 2016,

di ben 20 milioni di euro, una cifra estremamente significativa, in qualche modo però sostituita dalla maggiore spesa relativa alle pensioni.

della creazione e del rafforzamento, a maggior ragione dopo il risultato del *referendum* costituzionale del 4 dicembre, di servizi comuni tra Camera e Senato. Sono molteplici i servizi...

C'è un tema di servizi comuni, che credo sia estremamente importante (potrebbero esserne citati diversi); questa è una direzione che va assolutamente coltivata e credo che questo debba essere un mandato che in qualche modo lasciamo

nella prossima legislatura, sul tema della *spending review* - mi rivolgo ai Questori - credo che si possa fare di più. Provo a spiegarlo. C'è un dubbio di fondo strutturazione, in particolare, del bilancio di previsione. Per chi ha avuto, nella sua vita professionale (come è capitato a me), modo di confrontarsi con bilanci di azienda e quindi con logiche di tipo budgetario, devo dire che i numeri, per come sono costruiti nel bilancio di previsione, mi hanno lasciato molto perplesso. Questa è sostanzialmente una spesa storica che galleggia anno su anno. Detto in altri termini, le ottimizzazioni e i risparmi che si ottengono ogni anno non sono consolidati,

2016 (miglioramento significativo). Uno si aspetterebbe un bilancio di previsione per il 2017 con una cifra pari a 1.847.000 oppure, in una logica di miglioramento, invece il *budget* o la spesa di previsione per il 2017 è pari a 3.164.000, che è esattamente il *budget* del 2016. Per cui, a fronte di un *budget* di 3.164.000, se ne sono spesi solo 1.847.000; quindi si è fatto un grande risparmio. In questo caso abbiamo una cifra che va in diminuzione. Prendiamo invece il capitolo

Anche qui ci si aspetterebbe un bilancio di previsione per il 2017 per questo capitolo intorno ai 4 milioni di euro; invece è esattamente uguale a quello del 2016: 6.220.000. Se

Ho provato, con i numeri, a spiegare quello che mi sembra un elemento centrale, soprattutto per rendere la *spending review* strutturale. Qui le strade sono due: o si costruiscono i bilanci di previsione tenendo conto dell'andamento dell'anno precedente oppure questo galleggiamento della spesa storica porta in alcuni casi a non rendersi conto delle inefficienze che ci sono all'interno di questi capitoli. L'altra scelta, che si può leggere in qualsiasi libro di economia aziendale, è quella del *budget* a base zero, cioè rimotivare ogni anno le spese di ogni singolo capitolo. Questa è la strada vera, se vogliamo apportare significativi risparmi e rendere la *spending review* strutturale. Altrimenti, questo gioco dei risparmi e questo modo di costruire i bilanci di previsione impedisce in realtà di controllare e di premiare, in alcuni casi, i responsabili dei servizi che fanno una politica di *budget*. Detto in altri termini, affidare ad un responsabile

Nonostante queste osservazioni, che sono più di prospettiva e in qualche modo sono una sorta di messaggio messo nella bottiglia per la prossima legislatura, il Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista voterà a favore del bilancio del Senato.

vorrei fare una premessa. È convinzione del nostro Gruppo che vi siano ancora significativi e ampi margini per la riduzione della spesa nel bilancio e quindi della dotazione che il Senato riceve dallo Stato. Vogliamo qui richiamare l'attenzione dell'Assemblea su tre questioni, a nostro avviso particolarmente importanti, per le quali il Movimento 5 Stelle lotta da anni, ma alle quali questa Assemblea e il Consiglio di Presidenza non hanno ad oggi ancora dato una risposta.

Il primo tema che vorrei sottoporre all'attenzione riguarda ancora una volta i vitalizi spettanti agli ex senatori. Sono quegli stessi vitalizi rispetto ai quali avete votato contro stamane, per non perdere qualche giornata di ferie o forse perché essi sono una vostra creazione, dalla quale fate fatica a liberarvi e a staccarvi. Ebbene, fin dal 2013, il Movimento 5 Stelle ha cercato con diverse proposte di giungere all'eliminazione di questo privilegio del tutto inaccettabile dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Già molti anni prima che nascesse la proposta di legge sulla rideterminazione dei vitalizi con il metodo contributivo, che è stata approvata dalla Camera dei deputati, il Movimento 5 Stelle in Senato, consapevole del fatto che la regolamentazione dei vitalizi necessita o meglio necessiterebbe - di una deliberazione del Consiglio di Presidenza, ha proposto diverse soluzioni, che vanno dalla soppressione *tout court*, all'applicazione di un contributo di solidarietà, fino al ricalcolo dei vitalizi con il metodo contributivo.

sintomatica dello scarso livello di trasparenza in cui versa purtroppo questa istituzione, è la mancata rendicontazione da parte dei senatori dei rimborsi spese, che mensilmente ricevono per l'esercizio del mandato di parlamentari. i rimborsi spese sono esenti da tassazione, come ha ricordato poc'anzi il mio collega, ai sensi dell'articolo 52 del testo unico sulle imposte sui redditi. riteniamo che la rendicontazione puntuale delle spese e la restituzione all'Amministrazione di quanto non rendicontato - e quindi non speso - sia necessaria per ragioni etiche, prima che politiche, anche perché in questa maniera otterremmo il risultato di riavvicinare i cittadini alle istituzioni. Eppure, tutte le nostre proposte in tal senso, anche oggi, sono state respinte da questa Infine, la terza questione che voglio sottoporvi riguarda il servizio di cassa del Senato della Repubblica e lo sportello interno, che dal 2003 è gestito dalla BNL. La convenzione con la BNL è scaduta nel 2009 ed è stata dapprima prorogata annualmente. Poi, nel novembre 2011, con delibera del Consiglio di Presidenza, l'Amministrazione è stata autorizzata a prorogare il rapporto con BNL per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio e per il perfezionamento della relativa convenzione. Ebbene, sono passati sei anni da quella delibera ancora l'Amministrazione non è stata in grado di completare l'*iter* per l'affidamento in concessione del servizio di cassa e per la gestione dello sportello interno. Prendo atto che un ordine del giorno presentato accolto: questa potrebbe essere finalmente la chiave di volta rispetto al problema. Tuttavia, sono passati sei anni: alla faccia dell'efficienza! Per tutte queste ragioni, anche quest'anno abbiamo proposto diversi ordini del giorno che, ancora una volta, il Partito Democratico e la maggioranza hanno deciso di bocciare. Vorrei ricordarne qualcuno. Avete detto «no»,

ma c'è un interesse pubblico che deve essere tutelato. L'ordine del giorno G23 è particolarmente interessante:

Lo stesso ordine del giorno nel 2016, poi, è stato effettivamente dichiarato inammissibile; nel 2017 è stato dichiarato inammissibile, nel 2018 forse sarà dichiarato nuovamente ammissibile.

di ben 83 milioni di euro nel relativo capitolo di spesa del bilancio. È opportuno che anche i senatori, una volta cessati dal mandato, contribuiscano al contenimento della spesa del Senato? Credo di sì.

Avevamo chiesto l'abolizione dell'assegno di fine mandato: noi lo abbiamo già rifiutato, perché crediamo sia un privilegio a cui la politica può rinunciare per dare un messaggio al Paese, un Paese dove ci sono oltre 8 milioni di poveri. Sarebbe stato un bel messaggio, ma anche in questo caso avete detto «no». Abbiamo chiesto la riduzione dell'indennità e la rendicontazione, lo chiediamo ogni anno. Abbiamo proposto di mettere un tetto all'indennità di 5.000 euro lordi: noi già lo facciamo,

la diaria. Anche a questo avete detto «no». Abbiamo chiesto il dimezzamento delle spese forfettarie generali: anche questo sarebbe stato un bel segnale da inviare al Paese. E poi, la rendicontazione delle spese,

il Senato si ostini, in maniera opposta e contraria, a non considerare questi che sono tutto sommato piccoli gesti ma che molto direbbero ai nostri cittadini rispetto alla volontà di significare veramente una diminuzione dei costi della politica e, soprattutto, dei politici. Abbiamo chiesto la rendicontazione delle spese per l'esercizio del mandato: è una questione di trasparenza. Ci avete detto di no. Mi avvio a concludere. Abbiamo chiesto la riduzione del 20 per cento dei contribuiti ai Gruppi, ci avete detto di no. Abbiamo chiesto la pubblicazione dei precedenti,

Abbiamo chiesto delle misure economiche per contrastare il trasformismo parlamentare andando a intervenire sul portafoglio, ma ci avete detto di no. Abbiamo chiesto la soppressione dei rimborsi spese di viaggio degli ex senatori, che sono state sì ridotte, ma continuano a pesare per 400.000 euro sul bilancio

svolti in quest'Aula dal senatore Colucci e dal sottoscritto, nei quali abbiamo sottolineato e apprezzato le dichiarazioni del presidente Tonini in apertura. Abbiamo approvato la relazione, il rendiconto e il bilancio preventivo presentati dai senatori Questori. Ribadiamo che è stato fatto un buon lavoro con correttezza e trasparenza. Abbiamo posto il problema degli investimenti, soprattutto dopo dopo che il popolo italiano ha riproposto il Senato come Camera Alta della nostra Repubblica, e quindi la necessità, per non declinare, di investire maggiormente in risorse umane e materiali. Per questi motivi, il Gruppo di Area Popolare-Centristi per l'Europa esprimerà convintamente un voto a favore.

il clima che si respira oggi, rispetto a quello di un anno fa, quando abbiamo approvato il rendiconto e la previsione per il 2016, è un clima diverso, che determina un Senato vivo, confermato dal voto dei cittadini, quindi ci mette in una prospettiva diversa rispetto a quella che abbiamo respirato negli anni passati. Riprendo una considerazione fatto dal senatore Questore De Poli. Un Senato più semplice, più veloce, più efficiente: questo è l'obiettivo che penso tutti dobbiamo condividere, in relazione al nostro ruolo di essere trasparenti, una casa di vetro per i cittadini. Vorrei evidenziare la coerenza del bilancio con il dichiarato obiettivo di contenimento programmatico della spesa, un fatto che si rileva molto facilmente dai conti.

Il Senato pesa per 180 milioni in meno sulle spalle dei cittadini: è un fatto importante che testimonia l'impegno di tutti.

Alle critiche voglio rispondere che questo Senato dimostra, in realtà, la sua capacità di contenere la spesa, di lavorare bene, di razionalizzare, di mettere in comune risorse con gli uffici della Camera, riuscendo a dare quel servizio ai cittadini che si chiama democrazia. Settant'anni fa molti noi non c'erano e non possono avere che la testimonianza del frutto di chi ha dato anche la vita per poter essere qui a parlare. vorrei evidenziare che sicuramente emerge un continuo processo di miglioramento dei conti, intrapreso in questa legislatura, e la minor spesa ha assunto cifre significative e importanti. È importante sottolineare - come ho detto all'inizio - la trasparenza dei conti, che denota la volontà di fare le cose per bene. È per questo che noi esprimeremo un voto favorevole sia sul rendiconto che

Signora Presidente, senatrici e senatori, il dibattito odierno sul rendiconto delle entrate e delle spese del Senato relative all'anno 2016 e sul progetto di bilancio interno per l'anno 2017 è stato, come al solito, un momento di apprezzabile confronto, in cui si sono potuti sviscerare aspetti tecnici, importanti e sensibili, per la verità toccando anche qualche inesattezza, come quella che il collega senatore Crimi ha riferito in merito alle erogazioni liberali e alle dichiarazioni dei redditi. Faccio solo presente che non c'è alcun accumulo di questi aspetti, in quanto correttamente

questo dimostra che, quando un'istituzione discute, come abbiamo fatto oggi e come ha potuto fare anche lei - non credo sia un problema replicare alle inesattezze - e si approva un bilancio, si compie non solo un atto formale, ma anche un vero e proprio confronto politico e si valorizza il ruolo dell'istituzione e del Parlamento. Oggi tutti abbiamo sottolineato il prezioso lavoro dei Questori, di cui andiamo orgogliosi per i risultati portati, che consente alla nostra Istituzione di porsi con l'importante risultato di un conseguimento di tagli significativi, che però non hanno fatto venir meno la qualità dei servizi erogati. Mi sembra molto importante che nell'attuale momento nel Paese si dia questo tipo di esempio. È vero quanto ha detto il presidente Tonini: si può

alle sinergie e sicuramente grazie all'innovazione dei processi. Non sarebbe però possibile farlo se non ci fosse un'elevata professionalità del personale coinvolto. Credo che sia giusto, allora, sottolineare come, accanto a ciascun numero, a ciascun taglio, vi sia la volontà di adeguamento e di miglioramento prima di tutto del personale e sicuramente anche dei senatori e del Collegio dei Questori. Credo che tra i dati colpiscano molto - è stato riportato da molteplici colleghi - sia il risparmio netto conseguito,

Sono risultati che vanno sottolineati con orgoglio e apprezzamento, figli - lo ricordiamo - di quella svolta che è stata data nel 2012

linea che avete portato avanti, che potremmo riassumere con la parola efficienza, ma hanno anche invitato a fare di più,

della limatura probabilmente ha toccato i suoi livelli possibili, quella del miglioramento dei servizi è ancora implementabile e migliorabile. Mi riferisco, in particolare, alla possibilità

sottolineando come il dato della trasparenza sia uno di quelli su cui possiamo migliorare. Penso - ad esempio - a rendere pubblici in tempo reale sul nostro sito tutti gli elementi del bilancio, corredandoli possibilmente di quanti più dettagli possibili, anche nella fase annuale di analisi. Quelli delineati sono soltanto alcuni dei possibili interventi per visionare e migliorare il funzionamento del Senato e, più in generale, delle istituzioni parlamentari. di un campo d'azione oltremodo necessario, tenuto conto dei numerosi sforzi e sacrifici che tutta la collettività nazionale è stata chiamata a mettere in atto negli ultimi anni. Al Collegio dei Questori, anche sulla spinta delle determinazioni che assumerà l'Assemblea del Senato, spetterà formulare nei prossimi mesi le proposte che illustrino il percorso e le iniziative per proseguire nel percorso di complessiva riorganizzazione delle nostre istituzioni parlamentari.

noti anche quei dati medi che consentano di fare un'analisi di questo importante settore e - perché no - magari traguardare anche la possibilità che l'ente pagatore e gestore delle pratiche amministrative possa essere l'Amministrazione stessa, senza nulla togliere al rapporto diretto, che naturalmente è tra senatore e collaboratore. In conclusione, avendo ricordato tutti gli elementi di successo della nostra istituzione, posso posso esprimere con chiarezza il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. A nome mio personale e sicuro di interpretare i sentimenti di tutti i senatori, voglio ringraziare il Collegio dei Questori, nominativamente i senatori questori De Poli, Malan e Bottici e i loro collaboratori,

Ringrazio, inoltre, il Segretario Generale, i Vice Segretari Generali e tutti i loro collaboratori, che contribuiscono a far andare avanti al meglio

al nostro esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. È iscritto a parlare il senatore Crosio.

Innanzitutto, c'è una stortura nell'impianto di questo provvedimento, perché vi è l'evidente mancanza

Ricordo a me stesso che il 30 giugno 2019 verrà abolito il cosiddetto servizio di maggior tutela, che riguarda - per chi ci ascolta - la questione della bolletta elettrica. Una cosa è certa: noi siamo per la liberalizzazione del mercato. Ma è altrettanto certo che consegneremo agli italiani una bolletta più salata, e in modo particolare anche perché

non si è fatto nulla in questa direzione. Noi avremmo gradito - e lo abbiamo anche consigliato nei vari passaggi del testo tra Camera e Senato - la possibilità di tutelare il contribuente attraverso un possibile servizio di salvaguardia che andava verso i cittadini. Avete varato delle misure per quanto riguarda - ad esempio - gli impianti fotovoltaici che sono sui tetti delle nostre case e che

ahimè - non hanno la certificazione che dovrebbero avere - ma lo avranno fatto a loro insaputa - e vedranno decurtato il contributo che veniva dallo Stato

e non ha un piano industriale serio. Voi continuate a pensare che dobbiamo reperire energia a minor costo per poterla vendere a minor costo quando invece, tendenzialmente, nei Paesi più evoluti, che negli

è frutto di una politica che guarda di più alle *lobby* e agli interessi personali e non guarda assolutamente agli interessi del cittadino. Signora Presidente, colleghi, intervengo in sostituzione del collega Gianni Girotto, che ha seguito attentamente tutto l'esame del provvedimento ma che, purtroppo, non può essere qui con noi in questi lavori d'Aula. Il Movimento 5 Stelle conferma la sua opinione rispetto al provvedimento in esame sul quale si è già espresso contrariamente. Ritiene che, nonostante il lungo esame, la maggioranza non abbia saputo ascoltare le esigenze e cogliere l'opportunità che consumatori e attività produttive delle diverse categorie attendevano. Nell'esame lampo della quarta lettura tenuta in 10a Commissione, seppur non ci sia stata data alcuna possibilità di intervenire per apportare alcuni miglioramenti, si è invece palesemente dimostrata la difficoltà del Governo a mantenere i cocci di una maggioranza che anche in questo provvedimento è riuscita a tenere grazie al soccorso "crocerossino" di Forza Italia in Commissione e all'ennesima fiducia posta dal Governo in Aula. Sia il soccorso crocerossino che la fiducia posta dal Governo non entrano nel merito dell'argomento. Sono stampella di un Governo che, seppur senza maggioranza, vuol mantenere il suo impegno per preservare e curare gli interessi di bottega di diverse categorie, con un grave danno per la competitività del Paese e la tutela dei consumatori, piuttosto che lasciare aperto il libero confronto per intervenire e aprire realmente verso la liberalizzazione. un comportamento che allontana la maggioranza del Parlamento - e l'espressione politica che in questo momento sta rappresentando - dalla difesa degli interessi collettivi, alimentando l'egoismo degli interessi particolari. Approfondisco questo aspetto ricordando in quest'Assemblea la riflessione tenuta da Luigi Einaudi in «Economia di concorrenza e capitalismo storico». Egli riteneva in sostanza di riflettere sempre sul fatto che «la pianta della concorrenza non nasce da sé, e non cresce da sola; non è un albero secolare che la tempesta furiosa non riesce a scuotere; è un arboscello delicato, il quale deve essere difeso con affetto contro le malattie dell'egoismo e degli interessi particolari, sostenuto attentamente contro i pericoli che da ogni parte lo minacciano sotto il firmamento economico». Con l'approvazione di queste disposizioni, la pianta della concorrenza, rappresentata da Einaudi nell'arboscello delicato, rischia di essere minacciata dalle malattie dell'egoismo e degli interessi particolari che questa maggioranza ancora una volta ha voluto garantire. Gli argomenti affrontati sono stati molti. Ci soffermeremo solamente su alcuni degli aspetti che riguardano il settore dell'energia, che il Movimento 5 Stelle ha ritenuto opportuno far emergere durante i lavori. Sono proposte che il Governo e la maggioranza hanno fatto cadere nel vuoto, perché avrebbero aperto realmente il mercato dell'energia alla liberalizzazione e scardinato il sistema centralizzato e oligopolistico Noi abbiamo chiesto cose semplici. Abbiamo chiesto di non ostacolare la rivoluzione energetica e i suoi benefici in atto. Abbiamo chiesto di dare a tutti l'opportunità di poter produrre, autoconsumare e vendere energia da fonte rinnovabile, come stabilito dalle direttive europee, disapplicate Continuare a ostacolare la creazione di questo modello energetico decentrato, rinnovabile ed efficiente non aiuta la salute, l'ambiente e l'economia del nostro Paese che, dopo aver investito massicciamente - anche commettendo errori sui meccanismi di incentivazione che che non vogliamo nascondere - e maturato importanti esperienze e professionalità, rischia ora di lasciarle nelle mani degli altri Paesi. Ricordiamo che le aperture del collega Tomaselli e gli ordini del giorno approvati sui sistemi di distribuzione chiusi sono apprezzabili, ma non hanno portato ancora alcun cambio di passo. Se avreste realmente voluto, potevate intanto convergere sulla nostra proposta. Ma evidentemente non avete il coraggio di mettervi contro la grande *lobby* della produzione di energia centralizzata. Nell'ambito del mercato elettrico dell'energia, uno dei temi che ha spinto il Governo a porre la fiducia, avete cambiato troppo spesso le carte in tavola, inseguendo principi e obiettivi diversi, tutti contro i consumatori. Ugualmente avete creato maggiori incertezze per i consumatori, rinviando a un decreto del Ministero dello sviluppo economico la sorte di 23 milioni di clienti che attualmente non sanno come e cosa potranno scegliere per la fornitura di energia dal momento in cui il cosiddetto mercato tutelato sarà abrogato. Su questo aspetto il Movimento 5 Stelle ha voluto tenere una posizione coerente senza farsi tirare la giacca ed evitando che i clienti incapaci di scegliersi un fornitore fossero dati in pasto nel cosiddetto mercato di salvaguardia, con un meccanismo attualmente difficile da decifrare. Il Movimento 5 Stelle presterà molta attenzione per evitare che milioni di consumatori vengano dati in pasto senza tutele ai pochi produttori e venditori di energia, per superare realmente l'oligopolio presente. Siamo contrari a spingere i consumatori nella salvaguardia, ma favorevoli a rendere la gestione per la loro fornitura non a un monopolista, ma a una pluralità di venditori. Anzi, crediamo che il monopolio di ENEL sulla distribuzione debba essere finalmente superato, così come sia necessario nazionalizzare la parte che riguarda la trasmissione dell'energia fatta da Terna. Sono temi che avremo sicuramente modo di riprendere. Sarebbe stato opportuno accompagnare il consumatore in un percorso di crescita capace di generare consapevolezza e orientamento. Conosciamo bene il mondo delle bollette illeggibili. L'unica cosa comprensibile nella lettura della bolletta è il conto totale da pagare. Sono difficili da comprendere i servizi e i costi delle bollette telefoniche, per la fornitura elettrica e di qualsiasi altro servizio. Avremmo dovuto dotare il consumatore di strumenti efficaci di difesa. Invece, continuerà a essere vessato dalle grandi compagnie e un'altra occasione sembra che andrà persa. la prima cosa che mi è venuta in mente è che ci vuole un bel coraggio a chiedere la fiducia su un provvedimento di questo tipo. Dopo tutto il tempo Dopo tutto il tempo in cui si è cercato di modificarlo e migliorarlo per dare risposte a una serie di categorie che chiedono risposte alla politica, oggi esaminiamo un provvedimento che - a nostro parere - fa praticamente acqua da tutte le parti.

il problema della sanità, che viene toccata in modo preponderante; il problema delle comunicazioni e dell'energia, di cui ha parlato benissimo il senatore Crosio,

con una lettera importante che è stata mandata a tutti i senatori e allo stesso ministro Franceschini. La lettera contiene le stesse perplessità che abbiamo e che avevamo noi. Mi riferisco innanzitutto all'innalzamento dell'età che un'opera deve avere per essere considerata bene culturale:

per quanto riguarda la cultura e poi alla fine scivolano in modo pesante e preponderante su iniziative di questo tipo. Peggio ancora, sempre per quanto riguarda i beni culturali, è la liberalizzazione dell'uscita definitiva dal territorio del nostro Paese di tutti i beni culturali che abbiano un valore economico autodichiarato inferiore ai 13.500 euro. Io ho in casa un'opera che vale milioni di euro, dichiaro che vale meno di 13.500 euro e la posso esportare. Signora Presidente,

Signora Presidente, colleghi, stiamo esaminando un provvedimento importante che aprirà alcuni settori economici a una maggiore concorrenza, la quale servirà da volano a una maggiore crescita economica. L'impegno era di varare una legge sulla concorrenza ogni anno, mentre ne approveremo una in tutta la legislatura. Spero, quindi, che la prossima legislatura riesca a mantenere la periodicità annuale. non desidero entrare nel dettaglio dei contenuti, in quanto già fatto egregiamente dai relatori. Segnalo solo alcuni spunti di riflessione. Bisogna continuare la lotta senza sosta alla concorrenza sleale di chi evade le tasse, di chi non rispetta le regole sul lavoro mettendo a rischio la vita dei lavoratori. Tanto si è fatto in questa legislatura, come - ad esempio - con la legge sul contrasto al caporalato, ma c'è ancora tanto da fare. Bisogna inoltre intervenire con regole antidumping a livello europeo affinché carenti condizioni lavorative penalizzanti i lavoratori e loro sindacati, addirittura il mancato rispetto dei diritti dell'uomo, l'assenza di protezione dell'ambiente non diano un ingiusto vantaggio competitivo a nazioni di più recente industrializzazione.

mi riferisco alla legge francese sul dovere di diligenza per le società multinazionali e al *modern slavery act* (legge sulle moderne forme di schiavitù) del Regno Unito. Questo nostro disegno di legge, insomma, è molto concentrato sulla concorrenza di tipo commerciale e meno su quella di tipo industriale. terzo spunto di riflessione aprendo il mercato, avrebbe abbassato i prezzi a beneficio dei consumatori sarebbe stata necessaria e opportuna. Magari si sarebbero potute prevedere norme di tutela per le farmacie nei piccoli centri, ma sarebbe stato opportuno aprire questo mercato. Non intervenire è stato un errore, una ingiustizia. Infine, il presente disegno di legge arriva alla sua approvazione definitiva dopo molti passaggi parlamentari, dopo periodi di stallo in Commissione, dopo trattative e forzature di cui si è saputo poco e immaginato molto. Sarebbe stata auspicabile più trasparenza; si sarebbe potuta cogliere l'occasione per introdurre norme per regolamentare l'attività dei portatori di interesse. Le interferenze di gruppi di pressione ci sono state e non vi sarebbe stato nulla di deprecabile in questo se ci fosse stata vera trasparenza. La regolamentazione dell'attività delle *lobby* è una esigenza sempre più sentita a tutti i livelli. Recentemente la Camera dei deputati ha introdotto un registro dei lobbisti e ha definito regole per l'accesso al Parlamento; molte Regioni hanno deliberato in tal senso e così pure alcuni Ministeri. Manca però una legge nazionale e questa è una grave carenza. presente disegno di legge ho provato a proporre come emendamento la proposta legislativa che, in Commissione affari costituzionali, è il testo base per regolamentare l'attività dei portatori di interessi. L'esito, purtroppo, è stato negativo. In conclusione, stiamo facendo un importante passo avanti,

quindi di un articolato abbastanza importante, abbondante direi, essendo 15 gli articoli.

un prezzo ragionevole per il consumatore. Ma già all'interno del mercato RC auto sappiamo benissimo che diverse volte l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha dovuto bacchettare, e quindi sanzionare, le imprese, perché facevano cartello tra loro. E da ultimo - guarda caso

il sistema RC auto in Italia: un sistema che doveva essere cambiato, un sistema che doveva essere rifatto totalmente da capo, perché non c'era concorrenza e quindi, e quindi, non essendoci concorrenza, i prezzi non erano ragionevoli. E, quando abbiamo cominciato a fare battaglia, abbiamo notato che le imprese, imprese, probabilmente per una situazione che in automatico è capitata quando siamo entrati e abbiamo cominciato a parlare proprio di RC auto e - guarda caso - forse una situazione di rischio è venuta meno,

Ma vacci in Europa, cara mia compagnia. Unipol e ANIA, che siete venute in Commissione, andate in Europa; andate a parlare in Europa e dite che in pratica in Italia una stessa persona, con la stessa età,

se parliamo di concorrenza, allora parliamo di aziende. Un'azienda che ha la sua attività in una zona,

Senato farete la stessa cosa che avete fatto fare all'RC auto equa. Qui in Senato probabilmente l'abrogazione dei vitalizi non avverrà.

tutti gli automobilisti che negli ultimi cinque anni non dichiarano sinistri - e ciò vuol dire che sono automobilisti virtuosi - va applicato il premio più basso del territorio nazionale. In tal

È mai possibile che vengano qui in Senato a dirci queste cose? E noi cosa facciamo? Anzi, non noi, ma voi cosa fate? Fate quello che vi hanno chiesto! È ovvio che poi vengono dei dubbi,

avete fatto un provvedimento che non servirà a nessuno.

«Legge annuale per il mercato e la concorrenza». Signor rappresentante del Governo, mi rivolgo a lei per capire come il Governo e il Parlamento dovrebbero tutelare i cittadini.

Voglio chiedere al rappresentante del Governo come possa l'Italia uscire da un momento di difficoltà se i due problemi che affliggono il Paese sono uno sotto il profilo economico e commerciale e l'altro sotto il profilo sanitario.

Quando perciò sento il collega parlare di tutela del cittadino, e però non riusciamo a fare queste riflessioni, che sono veramente pesanti, credo stiamo parlando di qualcosa di astratto e sicuramente non possiamo offrire nessun tipo di garanzia.

previsto una tutela per il cittadino distinguendo quelle banche che in questo momento stanno sotto un'unica capanna e agiscono in un modo molto scorretto o poco ortodosso nei confronti dei cittadini.

più possibilità ai parlamentari di intervenire, sviscerare, emendare e creare qualcosa di più concreto nell'interesse del Paese. Spero per il futuro che il vostro Governo possa cambiare indirizzo, per il tempo che resta, e avere un rapporto diverso con i parlamentari all'interno di quest'Aula.

seppure arrivato alle battute finali, ha dimostrato tutta l'inadeguatezza dello strumento di una legge annuale per la concorrenza. Ciò, essenzialmente, per due motivi: il è che sono serviti quasi tre anni per completare una legge che dovrebbe essere, appunto, annuale; il secondo, come giustamente sottolineato dal presidente Mucchetti in Commissione industria lo scorso 27 luglio, soprattutto per le incertezze del Governo. Imputabile al Governo è soprattutto l'eccessiva vastità del testo in discussione: tante materie, tanti settori coinvolti che hanno prodotto però, al dunque, un risultato scarso per una felice apertura alla concorrenza dei mercati. La legge per la concorrenza si è trasformata, da provvedimento volto a liberalizzare, in un grande calderone che, più che aprire alla concorrenza in diversi settori, cerca di difendere maldestramente i consumatori e proteggere alcune categorie. Possiamo ravvisare, qua e là, qualche intervento normativo su alcuni settori, ma si fa fatica addirittura a definirlo un disegno di legge sulla concorrenza. Del resto, il testo che discutiamo nasce dalla fusione del testo originario, presentato dal Governo Renzi, costituito da 32 articoli, con altre sette proposte di legge concernenti l'assicurazione obbligatoria auto e natanti. Questo non è il concetto di concorrenza che ci è propria, e non lo è nemmeno per l'Autorità garante, che ha chiesto interventi normativi diretti a rimuovere i colli di bottiglia e gli ostacoli che bloccano lo sviluppo dell'economia e impediscono al mercato concorrenziale di produrre i suoi effetti, in termini di efficienza e innovazione. Il risultato è un mostro, non a tre teste, ma a 192 teste, che, come spesso accade, accarezza tutte le possibili discipline legate alla concorrenza, senza mai trattarle a fondo. Da questa storia possiamo trarre un insegnamento per il futuro. Se la legge vuole mantenere la sua cadenza annuale, dovrà essere snella e coinvolgere due o tre settori da liberalizzare ogni anno, con interventi chirurgici, capaci di coinvolgere, fin da subito, tutti gli

come altri Paesi hanno regolato i settori in esame e come il processo di apertura alla concorrenza si è svolto nel tempo. Ciò può aiutare un Paese tendenzialmente corporativo come l'Italia ad aprirsi gradualmente a maggiori livelli di concorrenza senza ritardi e senza traumi sociali. Questo approccio vale anche per le categorie professionali, settore notevolmente coinvolto dal provvedimento. Sulle professioni si sarebbe dovuto operare in modo da tutelare maggiormente l'utente, semplificare, sburocratizzare. Ma l'evidente e l'utile è naufragato nel caos delle mezze scelte e delle soluzioni di compromesso: i commi 142 e 154 disciplinano, rispettivamente, l'esercizio della professione forense e di quella odontoiatrica in forma societaria e sono disposizioni evidentemente contraddittorie. Se infatti per le società, anche a scopo di lucro, costituite da avvocati è obbligatorio che due terzi dei membri siano avvocati iscritti all'Albo, per le società che gestiscono studi odontoiatrici un mio emendamento avente il medesimo contenuto è stato più volte respinto. Voglio sperare che la spiegazione non sia che le cause di tribunale necessitano di professionalità certificata da un albo e le cure odontoiatriche no, perché forse al Governo è sfuggito che il "tre per due" è un'offerta commerciale che poco si addice ad un bene e un diritto costituzionalmente tutelato come la salute. Del resto, sappiamo bene che nel nostro Paese, grazie alla cosiddetta legge Bersani, ai liberi professionisti, sulle cui spalle pesa realmente la sconsiderata scelta della politica di non essere né liberista né statalista, ma irresponsabile e ridondante, non si riconosce nemmeno un equo compenso per il loro lavoro. Questo provvedimento non ha avuto il coraggio di recepire le molte richieste del mondo professionale, e addirittura le proposte di legge presentate, tra cui una anche a mia firma, che reintroduce l'equo compenso per i professionisti. Il risultato è che gli avvocati hanno un tariffario non perché venga riconosciuto un valore al loro operato, ma perché ad un altro potere dello Stato, la magistratura, offre una tabellina per decidere sulle spese di giudizio. Ci sono, in alternativa, schiere di architetti, geometri, commercialisti, ingegneri, medici, che sono costretti talora a lavorare quasi in rimessa per riuscire a stare sul mercato. Il tutto a svantaggio dei consumatori, che si trovano trovano davanti un mercato dove lo strillone più forte si accaparra il cliente, indipendentemente dalla qualità del servizio che rende. Un po' come accade in politica, dove ultimamente chi più urla, più viene creduto. Da ultimo, qualora ci fosse ancora la necessità di dimostrare che per il Governo i professionisti si dividono in serie A e B, come le squadre di calcio, è per me assolutamente inconcepibile che la liberalizzazione della professione notarile passi attraverso una riduzione del numero di abitanti (da 7.000 a 5.000) per ogni notaio e non attraverso un'omologazione della disciplina di questi ultimi a quella degli altri professionisti, rendendo possibile l'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale. In un'ottica concorrenziale e di snellimento delle procedure, nonché in coerenza con l'indirizzo normativo comunitario, che investe il provvedimento stesso, avevo avanzato delle proposte di modifica volte a favorire l'allargamento ai professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge n. 4 del 2013, in primo luogo alla platea dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità e, in secondo luogo, a quella dei soggetti che possono rappresentare il contribuente nei contenzioso tributario, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato la loro assistenza (il tutto analogamente a quanto di recente statuito con il decreto-legge n. 193 del 2016). Trattasi infatti di soggetti già autorizzati quali intermediari fiscali, nonché abilitati a rappresentare e assistere i contribuenti dinanzi agli uffici dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della avevano tutte l'obiettivo di garantire la tutela del consumatore attraverso la valorizzazione dei percorsi di qualificazione e certificazione dei professionisti *ex* legge n. 4 del 2013, nonché il superamento delle restrizioni per lo svolgimento di un'attività per la quale non si ravvisano esigenze di interesse generale di carattere ostativo all'apertura della concorrenza. Proposte che, oltre a non gravare sul bilancio dello Stato, in quanto non comportavano oneri aggiuntivi, avrebbero ridotto al contempo i costi e aumentato i vantaggi per i contribuenti e per le imprese, che avrebbero potuto avvalersi della professionalità di soggetti che abitualmente colloquiano con l'amministrazione finanziaria. Scorrendo il disegno di legge, poi, si intercetta un'altra delle anomalie tutte italiane, le parafarmacie, sulle quali, si sa, il vero soggetto che guadagna sono i grandi gruppi economici della distribuzione, che attraverso queste forme "né carne, né pesce" possono inserire il loro *business* nel diritto fondamentale della salute. Liberalizzare il settore delle farmacie non vuole dire dilatare a seconda delle necessità i farmaci che possono o non possono essere distribuiti o apparentemente meno spendere per poi, in realtà, più spendere. Liberalizzare coscientemente vuol dire passare da un criterio di «massimo numero» di farmacie per abitante a un criterio di «giusto servizio», così da fondere due necessità: la diffusione capillare sul territorio nazionale dei presidi sanitari per eccellenza e le legittime richieste dei nuovi operatori entranti, evitando soluzioni farlocche e insoddisfacenti che aprono a più gravosi problemi. RI))*. Signora Presidente, colleghi, siamo arrivati alla fine di un percorso lungo e carico di ostacoli, che ha impegnato il Parlamento e, in particolare, il Senato per ben due anni. Il disegno di legge per la promozione e lo sviluppo della concorrenza, presentato dal Governo il 3 aprile 2015, sta per divenire legge, un risultato che in realtà assomiglia più a un punto di inizio che a un traguardo, soprattutto in ragione delle tante polemiche che hanno caratterizzato il suo *iter* legislativo. Prima di condividere alcune riflessioni, desidero ringraziare il presidente della Commissione industria, il senatore Massimo Mucchetti, e i relatori, i senatori Luigi Marino e Tomaselli, per il modo con cui hanno gestito l'*iter* di questo provvedimento; per aver difeso l'autonomia del Senato da ingerenze esterne e, soprattutto, dalle interferenze del Governo e delle segreterie dei partiti. Abbiamo dovuto prendere decisioni non sempre scontate, sapendo che le aspettative su questo provvedimento erano tante e diversificate. E il peso di questa responsabilità si e avvertito da subito, motivo per cui non è stato sempre facile trovare un punto di equilibrio in merito alle singole disposizioni, ma anche nella scelta delle materie da includere. In questo senso, le critiche che sono state mosse al Senato in merito alla lentezza della discussione e alla scelta di aver introdotto articoli che non erano presenti nel testo presentato dal Governo, sono infondate. Indubbiamente i tempi potevano essere minori, tuttavia i ritardi che si sono accumulati non sono in alcun modo imputabili all'azione del Senato, ma sono stati voluti dal Governo anche in ragione di contrasti interni alla maggioranza. A cominciare dallo stop richiesto con l'approssimarsi delle elezioni amministrative del 2015, alla richiesta di sospensione dei lavori per permettere l'avvicendamento tra il ministro Guidi e il ministro Calenda, alla sospensione voluta da Palazzo Chigi in vista della campagna elettorale per il *referendum* dello scorso dicembre. Tuttavia, la soddisfazione di arrivare alle battute finali del provvedimento in esame è mitigata dall'amarezza dall'amarezza determinata da scelte politiche che hanno messo il Senato davanti a un vero e proprio *Diktat*, senza alcun margine di trattativa, ma con un invito implicito a prendere o lasciare, che non fa onore alle Assemblee legislative. Lo scorso aprile è stato chiesto al Senato di fare un passo indietro per garantire l'approvazione del provvedimento in esame entro la fine della legislatura, nonostante vi fossero ancora i margini per migliorare alcune disposizioni. Davanti all'eventualità di buttare al vento il lavoro di due anni, il buon senso ci ha persuasi a prendere la decisione migliore, ma non quella più funzionale per la realizzazione di questo progetto. Eppure, quest'accordo è stato inspiegabilmente infranto durante il passaggio alla Camera dei deputati, mettendo la parola fine al percorso condiviso che era stato deciso precedentemente. Tra l'altro, le modifiche decise dai colleghi deputati presentano delle criticità evidenti che hanno peggiorato il testo approvato dal Senato. è un esempio la scelta dei colleghi deputati di eliminare la norma che aveva introdotto dei vincoli per le imprese che operano nel settore dei *call center*, come l'obbligo per gli operatori di comunicare i dati identificativi del soggetto committente e lo scopo commerciale del contatto, ma anche il divieto di offrire servizi in abbonamento senza il previo consenso, espresso e documentato. una disposizione che poteva rappresentare un primo passo per regolare un settore che manifesta delle evidenti carenze. Al riguardo, ringrazio il Governo per aver accolto, seppur con modifiche, un mio ordine del giorno, volto proprio a concludere, nei pochi mesi che ci separano dalla fine della legislatura, l'*iter* dei disegni di legge che modificano il Registro pubblico delle opposizioni. un'apertura da parte dell'Esecutivo che dimostra quanto l'emendamento abrogato alla Camera dei deputati non sia in linea con le attuali sensibilità politiche. Anche in questo caso, però, le ragioni della politica hanno prevalso sulle questioni di merito, poiché in gioco in questo momento c'è la credibilità del Senato e del Paese. Da domani, tuttavia, l'impegno dovrà essere quello di considerare la legge sulla concorrenza un provvedimento che deve essere approvato a cadenza annuale. significa, quindi, abbandonare la cattiva abitudine di inserire sporadiche norme all'interno dei più disparati provvedimenti, senza una visione d'insieme, per emancipare il Paese dai veti incrociati che hanno fino ad oggi mantenuto l'Italia sempre un passo indietro rispetto al resto d'Europa. L'attenzione del legislatore, infatti, non sarà tanto concentrata sull'azione delle *lobby* che cercano di conservare i loro spazi d'azione, quanto dalle novità che arriveranno dal diritto europeo. Sul fronte nazionale, in particolare, sarà importante monitorare la normativa degli appalti pubblici, che si basa proprio sul principio della leale concorrenza. È opinione diffusa che il sistema delle soglie comunitarie nelle procedure di affidamento rappresenti un impedimento per il nostro apparato imprenditoriale, basato per il 90 per cento su piccole e medie imprese. Si tratta di un effetto negativo che, senza correttivi, penalizzerà soprattutto il Mezzogiorno, che rispetto ad altre parti del Paese ha una maggiore percentuale di imprese di piccole dimensioni. Sarà sempre di più l'Europa a costringerci a rivoluzionare la nostra concezione di concorrenza, rivedendo i dettami del nostro mercato interno, che dovranno essere monitorati per non arrecare danno all'economia interna. Nelle ultime settimane si sono sollevate accese polemiche in merito alla ratifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Canada, il cosiddetto CETA, soprattutto perché molti operatori economici ritengono alcune sue norme penalizzanti nei confronti del nostro *made in Italy*, da sempre protagonista dell'economia italiana. Inoltre, è in corso alla Camera l'*iter* sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri i necessari poteri per raggiungere gli obiettivi loro assegnati. Una riforma che è destinata a modificare le dinamiche tra Parlamento e *authority*, con una possibile riconfigurazione di competenze che potrebbe incidere anche sull'attuazione della legge annuale per la concorrenza. Elementi, questi, che il legislatore deve tener presenti, accompagnando i cambiamenti in quelle realtà nazionali e locali che per decenni sono state soggette alle regole di un mercato chiuso. Guidare le nostre imprese all'interno di nuovi scenari europei, attraverso norme quadro e leggi che prevedano un giusto periodo di transizione, dovrà essere un imperativo. In altre parole, è necessario che non si ripetano situazioni come quelle che hanno coinvolto il servizio dei taxi. L'Italia non può indugiare oltre per essere competitiva, credibile e affidabile nell'ambito dell'economia interna, ma anche per attrarre investitori stranieri. L'approvazione della legge sulla concorrenza era una tappa imprescindibile e a questo Parlamento va dato il merito di aver raggiunto questo obiettivo. Adesso siamo sulla strada giusta, non ci resta che percorrerla con senso di responsabilità. Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, anch'io, come molti in quest'Aula, ho provato disagio per i lunghissimi tempi di approvazione di questo provvedimento. Certo, è incredibile che un provvedimento di tale importanza strategica sia ancora qui, nel rimpallo tra i due rami del Parlamento, ma è anche vero che le questioni toccate sono articolate, complesse e che a volte si basano sull'equilibrio molto sottile tra il combattere le rendite senza per questo proibire la possibilità di profitto, come ha ricordato bene il relatore Luigi Marino. Questo voto non scioglie tutti i nodi del provvedimento, a cominciare dal fatto che alcune misure erano state pensate in un quadro che adesso è mutato. Presto dovremo rimettere mano ad alcuni elementi contenuti nel testo per andare verso una maggiore Intanto salutiamo però come un fatto positivo la sua approvazione, perché ci sono norme importanti, norme a lungo attese dai diversi ambiti economici che ne sono interessati. La concorrenza, quando corretta, stimola il confronto e porta al miglioramento dell'offerta. Come autonomisti, abbiamo sempre sottolineato la necessità di iniziative volte a snellire il quadro burocratico, in grado di premiare il merito e favorire la competitività, norme in grado di valorizzare le potenzialità del nostro sistema produttivo, che possano stimolare l'innovazione di processo e di prodotto, ma anche norme, soprattutto in quei mercati dove vi può essere la tendenza delle grandi corporazioni a determinare le regole d'ingaggio, in grado di tutelare le piccole realtà, quando sono di nicchia e producono qualità. Un equilibrio che va ricercato, anche rispetto all'interesse del consumatore. Ne è un esempio il fatto di aver scongiurato il rischio che siano le assicurazioni a scegliere i carrozzieri in caso di incidente. Il rischio, come è stato spiegato più volte in questi mesi, è che le prime arrivassero a stabilire prezzi e modalità lavorative delle seconde, diventandone quasi dei proprietari-ombra. Tra le altre norme positive ci sono quelle legate alle *smart city*, ad una maggiore trasparenza delle compagnie telefoniche, al mondo degli agrotecnici che hanno salutato positivamente le misure sul rafforzamento dello strumento societario per l'esercizio della professione. Vorrei poi menzionare un mio emendamento che dà la possibilità alle imprese che esercitano attività di trasporto-persone mediante autobus di utilizzare in locazione i veicoli di proprietà di un'altra impresa. Con questa misura le imprese iscritte al Registro elettronico nazionale potranno ottimizzare le risorse, favorendo un servizio più elastico, un mercato più dinamico. Sono solo degli esempi, ma credo rendano bene gli aspetti positivi, alcuni dei quali attesi dagli operatori del settore. Avevo poi presentato un emendamento sull'IVA telematica, che a mio avviso era molto importante, ma che purtroppo non è stato accolto. È stato invece un errore della Camera sopprimere la norma del codice delle assicurazioni private, precedentemente introdotta in Senato, che prevedeva che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia alla loro scadenza non potessero essere rinnovate tacitamente. Il collega Berger nelle dichiarazioni di voto domani farà un quadro complessivo dei miglioramenti che sono stati introdotti grazie ai lavoro del nostro Gruppo, a cominciare da quelli che vanno incontro ai bisogni dei territori e dell'economia di montagna, e sul quale mi sento anch'io di ringraziare il relatore Luigi Marino, il sottosegretario Gentile, i componenti della Commissione per il lungo lavoro, attento e puntuale, che si è svolto in Commissione. Da ultimo voglio ricordare il nostro ordine del giorno sulla questione legata al commercio parallelo dei farmaci; una pratica legale, con un fatturato di svariati milioni di euro l'anno, ma che rischia di creare problemi di disponibilità dei farmaci, soprattutto per quelli di classe A, A, tema su cui il Ministero della salute era già intervenuto in passato ma che non è stato ancora del tutto risolto. Per questo il mio auspicio è che, anche sulla scorta dell'accoglimento dell'ordine del giorno, vengano messe in campo iniziative atte a prevenire efficacemente stati di carenza o indisponibilità, anche temporanea, di alcuni medicinali essenziali sul territorio nazionale imputabili, direttamente o indirettamente alla pratica dell'esportazione parallela. È un tema importante, sul quale sarà necessario intervenire quanto prima per garantire la piena accessibilità ai farmaci e il diritto alle cure.

come il ministro Franceschini avesse potuto permettere l'inserimento del comma 176 in questo disegno di legge sulla concorrenza, che poi è diventato un articolone unico. Io, invece, non mi stupisco affatto, perché il comma 176 sulla circolazione dei nostri beni di interesse culturale all'estero è il degno epilogo di un film dell'orrore i cui sceneggiatori sono la premiata ditta Franceschini- Renzi-Madia. Il tutto nasce, con quel provvedimento d'avanguardia, il cosiddetto sblocca Italia, poi ribattezzato giustamente rottama Italia; del resto, lo ha voluto fortemente il rottamatore che finirà rottamato. Poi abbiamo avuto la riforma del Ministero, poi la legge delega Madia sul riordino della pubblica amministrazione, che ha visto questa bella norma sul silenzio-assenso e poi anche le Soprintendenze sono state poste sotto il commissariamento della prefettura. Ancora, abbiamo avuto il disegno di legge sui centri storici e il correttivo del codice degli appalti. Se non cambia qualcosa, avremo il disegno di legge di riforma della normativa sui parchi e, finalmente, arriviamo a questo comma 176 del disegno di legge sulla concorrenza. Tutto questo perché noi dovremmo essere garanti dell'articolo 9 della nostra carta costituzionale. Bravi noi: anzi, bravi voi. Questo comma 176 maschera una finta semplificazione aprendo l'autostrada per i beni di interesse culturale, che potranno allegramente uscire dall'Italia, con grande gaudio dei mercanti d'arte poco virtuosi, di tutti coloro che si sono dedicati a vario titolo all'esportazione

Come funzionava fino ad oggi? Gli uffici di esportazione del Ministero svolgevano (e in teoria svolgerebbero ancora) un controllo preventivo sulle cose suscettibili di essere beni di interesse culturale. I requisiti per il passaggio obbligatorio negli uffici di esportazione per l'uscita definitiva,

fossero stati eseguiti da oltre cinquant'anni. Cosa cambia, invece? L'innalzamento della soglia da cinquanta a settanta anni e l'introduzione di una soglia di valore economico.

Sul valore venale che viene introdotto come parametro per definire l'interesse culturale di un bene ci sarebbe da strapparsi i capelli, perché è una cosa sconcertante. Che cosa facciamo il valore culturale di una cosa con la sua quotazione, ma sappiamo bene che il valore culturale, a differenza di una quotazione, non è un valore ondivago che sottostà alle leggi del mercato, né un valore che per sua natura può essere mutevole o cambiare di luogo in luogo. Il valore culturale di un bene dovrebbe essere sganciato da tutti questi fattori variabili. Invece no: decidiamo che valore culturale di un bene d'ora in poi sarà assimilabile al suo valore di mercato. Bravissimi voi! Quindi, come giustamente ricordava un collega, tutte le opere prodotte tra il 1947 e il 1967 non saranno sottoposte al vaglio obbligatorio degli Uffici esportazione. E qui sono già stati citati illustri autori che hanno dato tanto e tanto lustro al nostro Paese:

perché non ci sono solo le tele. A proposito dell'autocertificazione essa è ammessa indipendentemente dall'età. Saranno liberi di uscire dal nostro Paese, senza il vaglio dell'Ufficio esportazione, tutte le opere di valore inferiore ai 13.500 euro.

a rispettare la norma stringente sul silenzio-assenso, perché se non rispetteranno i termini prescritti, che sono stati dimezzati, vedranno partire opere, con devastazione del nostro paesaggio, senza colpo ferire. I soprintendenti saranno tutti impegnati a salvare il nostro paesaggio e il nostro patrimonio e dovranno anche prendersi la briga di andare a consultare, *una tantum*, questo registro informatico tenuto dei mercanti d'arte, chiedere di poter visionare il bene sospetto e verificare così l'autocertificazione. C'è di più:

senza la preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, ossia il prefetto. Con una leggina, il decreto legislativo n. 222 del novembre 2016, abbiamo abrogato l'articolo 126, di fatto abrogando l'obbligo di questa dichiarazione.

depotenziato uno strumento. Chiediamo quindi ai mercanti d'arte di tenere uno strumento, senza alcun obbligo di fare alcuna dichiarazione, né all'autorità preposta alla pubblica sicurezza, ossia al prefetto, né al soprintendente, perché sarà il soprintendente a doversi prendere la briga di effettuare eventuali controlli su controlli su tutti i mercanti d'arte e tutti quelli che commerciano i libri antichi e manoscritti. Ci siamo già dimenticati, infatti, della favolosa vicenda che ha interessato la Biblioteca dei Girolamini di Napoli. Ci siamo già dimenticati di tutta quella marea di manoscritti trafugati, vicenda per la quale abbiamo anche un noto esponente politico che in questo momento non è più tra noi, ma altrove, mi pare a Parma. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ecco, ci siamo dimenticati di tutte queste cose, perché la nostra memoria corta è proporzionale al nostro interesse per la tutela del nostro patrimonio artistico e culturale in questo Paese

C'è scritto che, secondo la nuova disposizione che si intende inserire all'articolo 10, anche gli oggetti di interesse archeologico non potranno essere vincolati se realizzati da artista ancora vivente. Ci metteremo tutti a fare delle belle sedute spiritiche e a richiamare questo artista vivente

e i settanta anni. Ancora una volta non è dato capire se per gli oggetti archeologici ci si intenda riferire all'epoca della scoperta o ad altro. Tutti questi potranno essere vincolati solo se di valore eccezionale non in sé, ma per l'integrità e la completezza del patrimonio nazionale, come se noi potessimo tranquillamente esportare tutte le cose ritrovate a Pompei perché, siccome non le abbiamo ritrovate nella loro completezza, verrebbero a perdere il loro valore eccezionale. Complimenti! In questa legislatura il ministro Franceschini e il Governo di cui fa parte saranno ricordati per lo scempio della tutela della tutela e della valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, credo che questa fiducia dia un po' il segno distintivo di un percorso accidentato di un provvedimento che ha impegnato

Grazie l'angolatura delle professioni, vedere questa particolarità e lo spazio che vi riserva il disegno di legge. Sicuramente il comparto è importante per il Paese due milioni di professionisti iscritti all'albo. Il comparto aiuta davvero a dare lavoro e contribuisce al PIL della nostra Italia. Il comparto ha avuto questo anno, da un lato, un riconoscimento importante con la legge sul lavoro autonomo e le deleghe nuove per le professioni, la semplificazione, qualche diritto riconosciuto e qualche passo importante. È per questo che vedo un po' distonico questo provvedimento. Esaminando ciò che

ma anche per l'impossibilità di compensare crediti e debiti con l'Agenzia delle entrate sotto i 5.000 euro; per il tema dell'equo compenso, una misura incompiuta. Dopo le "lenzuolate" del 2006 di Bersani, è un tema che viene posto con forza

il rispetto della funzione dei professionisti all'interno delle società di capitali. Non c'è un solo riferimento a un tutore deontologico dell'attività del professionista rispetto al capitale che giustamente o ingiustamente - non voglio affrontare questo tema - farà il suo lavoro, quello cioè di portare un utile all'azienda o una positività nel bilancio.

presente capitale esterno che è stato regolarizzato dal presente disegno di legge; avremo una diminuzione minima del bacino di utenza dei notai; abbiamo sicuramente situazioni non chiare per quanto riguarda l'ultrattività delle polizze, che saranno un ulteriore costo a carico dei professionisti. Io vorrei dire che se davvero avessimo voluto varare un provvedimento sulla concorrenza avremmo dovuto cercare di raddrizzare un po' il tiro, evitando di adottare un provvedimento che vuole affrontare tutti i temi per poi non affrontarne più, perché è impossibile seguire puntualmente l'evoluzione di una norma che contiene un po' di tutto. Ovviamente in questo caso non ha giovato il tempo, che ci ha fatto prendere e riprendere l'argomento tante volte e quindi perdere anche l'unità di azione. Vorrei tuttavia dire che, se davvero vogliamo dare una mano ai professionisti, con il provvedimento in esame non otterremo nulla, anzi avremo la mortificazione di chi tutti giorni, anche facendo fatica in questi anni, è riuscito a dare un contributo a questo Paese in termini di posti di lavoro e di PIL. Sicuramente su queste norme bisognerà ritornare,

Parto dall'assunto che non è più accettabile che ogni dieci anni cittadini, associazioni e sindaci della Val di Sangro (che è l'area industriale più grande d'Abruzzo) debbano combattere una battaglia già più volte vinta in passato. Quest'area ha già visto per ben due volte la bocciatura di progetti simili da parte del comitato di VIA regionale, ciononostante le imprese petrolifere si ostinano ancora. Reputo inammissibile che, nonostante le criticità di quell'area siano immutate e addirittura evidenti fin dal 1969, gruppi petroliferi internazionali si ostinino a presentare istanze per lo sfruttamento di questi siti. Quell'area ha il più grande giacimento su terraferma accertato in Italia, ma contestualmente è anche il più problematico. Nel 2009 la società Forest Oil SpA forestale presentò un'istanza di concessione, poi la Regione Abruzzo si si espresse con parere negativo sia nel 2012 che nel 2013, poi nel 2015 arrivò addirittura la bocciatura del Consiglio di Stato grazie ai ricorrenti del Comitato di cittadini Gestione partecipata del territorio del

di parere da parte del comitato di VIA nazionale, come se l'accertata e perpetua fragilità del territorio non fosse acclarata. La subsidenza potrebbe comportare seri problemi di tenuta della diga del Lago di Bomba e per questo, applicando il principio di precauzione, il comitato di VIA della Regione allora bocciò il progetto ora inopinatamente riproposto al livello governativo nazionale. Quel territorio deve essere escluso una volte per tutte dall'elenco dei giacimenti sfruttabili. I petrolieri della CMI Energia hanno recentemente depositato al Ministero ulteriori documenti; quindi a breve ci sarà la decisione della commissione VIA nazionale, a cui seguirà il decreto interministeriale. Ci dobbiamo domandare: come mai temi come la sismicità indotta, la subsidenza, la questione della sentenza del Consiglio di Stato e tante altre oggettive criticità sollevate in maniera approfondita vengono sottovalutate? L'ultimo provvedimento della riforma della VIA non fa che aumentare le preoccupazioni, visto che prevede che si possa andare avanti con il progetto, se il Ministero acconsente, anche in caso di bocciatura del provvedimento di VIA da parte della magistratura amministrativa. Quindi un parere favorevole, signora Presidente, del Ministero a questo progetto sarebbe davvero un colpo durissimo e inaccettabile per un'intera parte della Regione Abruzzo. La ringrazio ancora per il tempo che Signora Presidente, intervengo per l'ennesima volta per sollecitare l'attivazione della Commissione d'inchiesta sulla ricostruzione dell'Aquila.

membri, l'articolo 8 del Regolamento del Senato dice: «Il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Regolamento». Regola l'attività di tutti i suoi organi. Qui c'è un'attività che non riesce ad essere consentita. Tra l'altro, nella scorsa legislatura,

nonostante tutte le sollecitazioni e a un giorno dalla chiusura per la pausa estiva, non abbiamo avuto né una seria presa di posizione, né una chiara informazione su quali sono i Gruppi che continuano a tenere bloccata una Commissione d'inchiesta utile, utile, necessaria, urgente e indifferibile.

a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali, adottata il 28 luglio 2017